*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio oggi ricordare brevemente un'esperienza che è stata fondamentale nella mia vita e in quella di molti colleghi parlamentari che oggi all'alba hanno rinnovato l'antica promessa collegandosi idealmente a tutti quelli che nel mondo condividono gli stessi valori. Infatti, il 1° agosto 2007 milioni di *scouts* di guide hanno celebrato in tutto il mondo l'alba di un nuovo secolo di scoutismo e questo avviene esattamente a cento anni dall'avvio del primo campo sperimentato da Robert Baden Powell sull'isola di Brownsea. È un'occasione irripetibile per mostrare la forza sociale e la grandezza dello scoutismo nel mondo, perché è il momento in cui tutti gli *scouts* e le guide si uniscono con spirito di amicizia e di pace, orgogliosi delle proprie radici culturali, consapevoli della modernità della proposta educativa. Il 2007, anno entro cui si stima che più di 500 milioni di uomini e di donne avranno pronunciato la promessa nel mondo, è un anno ricco di eventi organizzati non solo per celebrare il passato, ma soprattutto per far conoscere la visione sul futuro di un movimento che continua ad essere vicino alle aspirazioni ed ai bisogni dei giovani che vivono in società in costante evoluzione. L'alba del centenario è il momento per ribadire con convinzione la priorità di movimento mondiale, nazionale e locale; è un giorno per dimostrare l'impegno attivo nel coinvolgere i giovani alla partecipazione nella società civile, nel favorire le relazioni paritetiche, nello stimolare a vivere l'ambiente in modo equilibrato e sostenibile, nel formare al volontariato e alla solidarietà, nel contribuire alla costruzione di un mondo migliore. *(Applausi dal

Presidente, lei mi ha ovviamente e autorevolmente anticipato. Ringrazio il senatore Tomassini di aver ricordato a tutti noi ciò che è avvenuto questa mattina in diretta mondiale alle ore 8, ringrazio il senatore De Angelis che era con me presente stamattina insieme al Presidente del Consiglio, ad altri Ministri della Repubblica e ad altri colleghi al Circo Massimo in questa occasione storica. Signor Presidente, molti senatori hanno sottoscritto, perché lei lo sappia, la partecipazione come soci fondatori all'Associazione parlamentari

tutte le istituzioni che avrebbero potuto essere interessate ad una azione diretta a bloccare questo sperpero di denaro pubblico.

Mi sono poi recato anche presso la procura di Santa Maria Capua Vetere al fine di far emergere quale fosse il tipo di gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

Ho denunciato anche la presenza di un presunto magistrato, ambientalista, il signor Tecce, che faceva da mediatore tra la camorra

su quelle stesse motivazioni, su quelle stesse constatazioni, su quelle stesse notizie fornite dal sottoscritto nel 2001, e successivamente,

e rendergli onore per tutto quello che ha dato alla cultura del Paese e di questo pianeta. Altri, più di me, sapranno semioticamente illustrare la grandezza di questo regista. Io lo voglio solo ricordare in uno dei suoi film meno riusciti - devo dire -, «Zabriskie Point», quando, in conclusione, Diana guarda la villa nel deserto e con gli occhi distrugge tutta l'inutilità di una società che aveva accumulato e non sapeva

Questo esito si è determinato per il combinarsi di tre fattori. Il primo è quello dell'esiguità del tempo a disposizione.

- sollevo tale questione perché vi sia una verifica del lavoro con l'altro ramo del Parlamento - che la Camera dei deputati ha impiegato 50 dei 60 giorni a disposizione

Il secondo fattore di difficoltà è quello relativo alla complessità ed alla eterogeneità delle norme contenute nel decreto e, ancora di più, nel disegno di legge di conversione, dopo le numerose modifiche introdotte dalla Camera. Naturalmente, caso è del tutto evidente che il carattere del decreto, una manovra espansiva, ha sollecitato l'introduzione nel decreto stesso di una serie di norme che erano in discussione nei due rami del Parlamento, avevano a che fare con misure di politica fiscale in particolare e si era colta l'occasione di questo veicolo per introdurre sul veicolo tutti i vagoni, per continuare con la metafora del treno, in quel momento oggetto di attenzione sia alla Camera sia al Senato.

assumere atteggiamenti tartufeschi - dalla perfetta consapevolezza della maggioranza e dell'opposizione della intenzione del Governo, dato l'incombere del «generale agosto», di apporre la questione di fiducia sulla legge al nostro esame. Posso quindi, signor Presidente, darle conto e dare conto all'Assemblea soltanto dell'andamento della discussione generale, in buona sostanza, che si è svolta in Commissione, nel corso della quale nel corso della quale sono state affrontate due questioni, negli interventi dell'opposizione, della maggioranza e del Governo, entrambe di grande rilevanza. La prima investe la scelta politica del Governo di realizzare immediatamente, a mezzo anno, un intervento espansivo che peggiora di quasi mezzo punto di prodotto interno lordo il dato dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni, così come si sarebbe determinato, prima del decreto, sulla base del tendenziale 2007 a legislazione vigente.

dello 0,4 per cento del PIL. La discussione su questo punto si è concentrata sulla scelta politica relativa all'opportunità o meno, sostenuta rispettivamente dalla maggioranza e dall'opposizione, di dar luogo a un intervento di questo tipo, in un contesto di crescita economica nel quale tradizionalmente l'adozione di una manovra prociclica come quella in esame è da sempre sottoposta a importanti valutazioni critiche.

dal bilancio a legislazione vigente, il quale però - qui c'è un punto assai delicato - non è stato ancora approvato dal Senato e dalla Camera, non è quindi una legge ma un disegno ma un disegno di legge. Sulla prima questione, quella relativa alla scelta politica di porre in essere una manovra espansiva a metà anno utilizzando le maggiori entrate cui ho fatto riferimento, si sono confrontate pozioni squisitamente politiche, che potranno emergere nel corso della discussione generale e che essendo posizioni politiche contrapposte naturalmente potranno risultare chiare a lei e ai colleghi nel corso della discussione che inizieremo tra qualche minuto.

rivolgendomi a lei, signor Presidente, e anche ai colleghi - ammesso che ce ne sia qualcuno interessato all'argomento La prima questione a proposito di copertura è, grosso modo, la seguente. È corretto sotto il profilo della legge di contabilità disporre l'utilizzo di maggiori entrate previste da un disegno di legge di assestamento che non è stato ancora approvato definitivamente dal Parlamento? L'opposizione nel corso di questo dibattito ha risposto a questa domanda con un rotondo no. L'articolo 11-*ter* della legge di contabilità richiede che per far fronte a nuovi oneri introdotti da nuova legislazione - è questo il caso - si provveda con risorse recate da nuove norme di entrata o di minore spesa, non da variazioni di previsione di entrata non ancora definitive e non ancora fissate in una legge perfettamente approvata. La legge di contabilità - è sempre l'opposizione che parla mio tramite - è norma attuativa dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e quindi prevale quindi prevale su qualsiasi disposizione della legge finanziaria in vigore, che, per quanto importante, è pur sempre una legge ordinaria e non una legge attuativa, come nel caso della legge di contabilità, della norma costituzionale. Questo - spero che i colleghi dell'opposizione me ne daranno atto - è stato il fulcro, naturalmente sviluppato con argomenti che adesso non posso riprendere, degli degli argomenti sviluppati dall'opposizione per sostenere la scorretta soluzione del problema della copertura finanziaria del decreto al nostro esame. La maggioranza non ha potuto e non ha voluto negare il fondamento di questa obiezione, ma le ha contrapposto un ragionamento incentrato sulla corretta applicazione, a suo dire naturalmente, dell'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria in vigore, quella del 2007. Le maggiori entrate - ha sostenuto la maggioranza - sono assolutamente certe e sono state utilizzate per coprire nuovi oneri solo per la parte delle stesse entrate maggiori a carattere strutturale, destinando, invece, la parte non strutturale di quelle maggiori entrate alla riduzione del livello dell'indebitamento, così come richiesto dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria. Quanto al riferimento al disegno di legge di assestamento - ha sostenuto sempre la maggioranza - ci sono precedenti importanti di comportamenti analoghi a quelli adottati in questo caso. In particolare, c'è quello relativo al settembre del 2000, quando effettivamente venne adottato un provvedimento a valer per i suoi aspetti di copertura su un miglioramento delle entrate non ancora perfettamente registrato dall'assestamento approvato, ma registrato soltanto attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di assestamento ancora da approvare da parte del Governo. Il confronto

a proposito della corretta copertura del provvedimento, a loro dire, ha finito per indurre la discussione a concentrarsi sulla valutazione circa il carattere strutturale o meno delle maggiori entrate. in particolare é stato indagato il tema di particolare delicatezza - che naturalmente viene affrontato in sede accademica, ma che qui ha immediate ricadute politiche politiche - del grado di elasticità delle entrate alla crescita del prodotto interno lordo. Il grado di elasticità

Si tratta di capire, attraverso lo studio del livello di elasticità, quali previsioni si possano fare in termini di entrate future, in presenza di aumenti del prodotto interno lordo più significativi rispetto a quelli che sono incorporati nelle previsioni che, quindi, hanno trovato attuazione nella valutazione nella valutazione delle entrate nel bilancio a legislazione vigente. Specificatamente - questo forse è un particolare che potrebbe interessare ai colleghi perché è un dato del tutto anomalo - si è rilevata l'assoluta anomalia del livello di elasticità delle entrate alla crescita del prodotto interno lordo registrato nel 2006. Il dato è veramente impressionante. Un ottimo studio del Servizio del bilancio della Camera e del Senato - approfitto per annunciare che per la prima volta i Servizi bilancio di Camera e Senato sul Documento di programmazione economico-finanziaria hanno prodotto un unico studio con le due firme,

come nel 2006 il livello di elasticità delle entrate, alla crescita del prodotto intorno lordo che oggi noi possiamo registrare (cioè come dato a consuntivo), é stato triplo rispetto rispetto a quello medio registrato nella serie storica ricavabile dalla serie storica degli anni precedenti. La serie storica degli anni precedenti produceva un livello di elasticità pari, grosso modo, a 0,9-1-1,1; il livello di elasticità delle entrate al prodotto interno lordo del 2006 è stato pari, signor Presidente, a 2,7, cioè esattamente tre volte il livello medio registrabile negli anni precedenti.

per forzare il dato delle previsioni di entrata, anche con riferimento al 2008, potremmo incorrere in errori di politica economica e di gestione della finanza pubblica particolarmente gravi, se non addirittura catastrofici. quindi assumere un atteggiamento di assoluta prudenza nella valutazione della previsione del livello di elasticità delle entrate del 2008 (e del 2007, per l'anno in corso) rispetto all'aumento del prodotto interno lordo, perché il dato del 2006, essendo certamente del tutto anomalo, andrà indagato. Voglio ricordare che alcuni degli errori più gravi di politica economica e di gestione della finanza pubblica commessi negli ultimi dieci anni

atteso del prodotto interno lordo. Spesso, vi è una sfasatura temporale tra i due fenomeni: la crescita del prodotto interno lordo, che sta alle spalle, viene proiettata passivamente nel futuro; su quella proiezione si costruiscono previsioni di entrata gonfiate e, sulla base di questo, si commettono errori di gestione della finanza pubblica particolarmente gravi. Questo è stato l'oggetto della discussione svolta in Commissione,

e anche per aver cancellato ogni tentazione tartufesca, come egli stesso ha voluto sottolineare. Questo mi pare il senso dell'intervento del senatore Calderoli. Ciò renderà più efficace la discussione, com'è stato evidenziato.

Va dato atto alla sua onestà intellettuale di aver riferito esattamente i termini con i quali in Commissione bilancio sono emerse questioni rilevanti,

all'interno del Governo e tra questo e la sua maggioranza, nel sottolineare la dichiarazione del sottosegretario Sartor in occasione della discussione sul DPEF. indicava una strada precisa al Governo, ossia perseguire gli obiettivi di *deficit* pubblico attraverso il contenimento della spesa primaria, contro una risoluzione - votata in quest'Aula dalla maggioranza - in cui si intravede, invece, la possibilità di aumentare ulteriormente la tassazione. Abbiamo registrato recentemente un altro segnale di stato di confusione mentale, attraverso la risoluzione approvata alla Camera dei deputati, che è a sua volta diversa da quella approvata qui in Senato; non si capisce quindi che cosa dovrà fare il Governo, se dovrà seguire le indicazioni del Senato o quelle della Camera. Ricordo in particolare che la risoluzione approvata dalla maggioranza alla Camera fa addirittura esplicito riferimento all'uso delle riserve della Banca d'Italia. È un ulteriore segno di stato di confusione mentale: riserve della Banca d'Italia, al di là del tema dell'autonomia della Banca d'Italia, non può ovviamente che essere un'operazione *una tantum* eventualmente essere utilizzate, non possono che andare a finanziare spese di investimento. Nulla hanno a che vedere, dunque, con il tema del contenimento della spesa corrente primaria. Bene, questo decreto, signor Presidente, è un'ulteriore clamorosa dimostrazione che quest'Aula tra oggi e domani vedrà, da parte della maggioranza e del Governo,

Il presidente Morando ha già indicato alcuni elementi emersi in Commissione bilancio ed è per questo che poniamo una pregiudiziale

33 è riportata una tabella in cui il Governo scrive che l'indebitamento netto tendenziale per il 2007 è pari al 2,1 Nelle righe successive scrive che l'effetto del decreto-legge al nostro esame sull'indebitamento netto è pari allo 0,4 e che pertanto il Governo pone per il 2007 un obiettivo, dopo il decreto, pari al 2,5 Signor Presidente, questo è un documento ufficiale del Governo e del Parlamento: in questo Documento il Governo dice che il decreto oggi in esame è totalmente finanziato con aumento di disavanzo.

il 2007 così recita: «Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 (...) sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale (...)». Ebbene, questo decreto non riduce l'indebitamento, anzi l'aumenta; non riduce la pressione fiscale, anzi l'aumenta, e aumenta la spesa pubblica corrente: esso è quindi incompatibile con il comma 4 della vostra legge finanziaria, che non mi risulta essere modificata. La terza motivazione è la seguente. Lo ha già detto in modo assolutamente ineccepibile il presidente Morando: questo decreto utilizza entrate emerse (che, come i colleghi sanno, rappresentano la controprova del falso in bilancio che avete commesso a dicembre), a dicembre), utilizza maggiori entrate prima che queste siano state iscritte a bilancio con il bilancio di assestamento. ore 10,37 di oggi, 1° agosto, le disponibilità in termini di entrate delle pubbliche amministrazioni iscritte a bilancio sono ancora pari a 703 miliardi di euro, che è il medesimo

formalmente non avete fatto emergere le entrate? L'aveste fatto a dicembre, quando ve lo avevo detto, sarebbe stato tutto perfettamente legale. Ma c'è di più, signor Presidente. Questo riguarda esclusivamente il 2007. il 2007. Circa l'effetto del decreto sul 2008 e sul 2009, nel decreto stesso viene detto che la copertura è data dai numeri scritti nel DPEF: non mi risulta che il Documento di programmazione economico-finanziaria sia una legge. Come si fa a dire che le maggiori spese indotte da questo decreto, a valere sul 2008 e sul 2009,

nel Documento di programmazione economico‑finanziaria, quando la legge di contabilità dice chiaramente che debbono essere coperti con i numeri scritti nelle leggi dello Stato, non nelle risoluzioni (peraltro contraddittorie) tra Governo e

relativamente ad una palese manovra di correzione a valere sul 2008 di 25 miliardi di euro. Se il Governo farà emergere i i 10-12 miliardi in più di entrate che ancora nasconde nei cassetti, comunque ci sarà bisogno di una manovra di almeno 15 miliardi di euro.

con un Governo che apporrà il voto di fiducia: un voto di fiducia per aumentare il *deficit* pubblico e continuare nella linea di non trasparenza, di non chiarezza del bilancio degli italiani. Dietro il suo scanno, signor c'è una frase di Vittorio Emanuele II. Quella frase fu scritta perché in quel momento l'Italia ascoltò un grido di dolore. Ebbene, mi rivolgo al Presidente della Repubblica, che ha controfirmato il decreto, e al presidente della Corte dei conti perché ascoltino almeno il grido di stupore con il quale in quest'Aula si assiste ad un delitto finanziario contro le leggi, contro le regole, contro una corretta contabilità, contro il buonsenso, contro gli organismi internazionali. Perché avviene questo? Perché avviene questo? Per dare qualche settimana di vacanza e aspettare a settembre un medico che certifichi la morte di questa maggioranza? *(Applausi dai Gruppi AN e

uno che riguarda il mancato rispetto dell'articolo 1 della legge di contabilità, l'altro per il contenuto proprio dell'articolato che riteniamo improvvido nell'utilizzazione dell'extragettito derivante dall'andamento tributario alle finanze dello Stato. Signor Presidente, l'articolo 1 di fatto riscrive una condizione ripetutamente inserita nella legge finanziaria e, in ultimo, al comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria 2007.

rispettando uno specifico comma della legge di contabilità, dove viene previsto che la legge finanziaria debba indicare altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio triennale non possa essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese, introduce...

(non permettendomi di parlare agli altri colleghi perché probabilmente quello che dico, anche se invitato a non fare polemica ma a collaborare da parte del ministro Visco, avrà dei contenuti di polemica) per non suscitare critiche mi permetterò di rivolgermi sempre e costantemente alla Presidenza, Presidenza, ma mi viene leggermente difficile - mi consentirà - poter argomentare se almeno lei, Presidente, non mi presta attenzione; capisco che è un compito difficile ma sa, lei è Presidente dell'Aula e oltre agli onori ci sono gli oneri: l'onere è quello magari di sentire me, ma cercherò di essere breve e di divertirla un po'.

Questo è possibile che sia sviluppato in filosofia, ma in matematica finanziaria il sillogismo finisce per diventare teorema e sappiamo che all'interno del teorema c'è la preposizione di base, cioè quella per cui per essere un teorema dimostrato ci vuole una condizione necessaria e sufficiente.

che la vecchia possa essere strega; condizione necessaria e sufficiente perché la vecchia sia strega è, non solo che abbia la scopa, ma che voli. Ora, il Governo la condizione necessaria per approvare è che ci siano i soldi: che ci siano i soldi lo sappiamo tutti, perché c'è l'extragettito, ma la condizione necessaria e sufficiente per prodursi una legge di spesa a legislazione vigente è che sia rispettata la legge di contabilità. Quindi, non è possibile soltanto che ci siano i soldi, ma che ci sia la condizione necessaria e sufficiente che i soldi ci siano e sia rispettata la legge.

perché sia testimoniato dall'opposizione - il cui compito ritengo sia questo - e si riesca ad indicare all'Aula, al Paese, agli altri parlamentari, a chi si occupa di contabilità dello Stato che il Governo si produce in una costante e continua violazione della legge di contabilità. Ne siamo stati testimoni ultimamente quando è stato votato il decreto per l'emergenza rifiuti, allorquando ha disposto una norma che era propedeutica a quello che sta avvenendo in quest'Aula, cioè

con una legge formale, che è la legge di assestamento, la quale è un bilancio in piccolo ma ha la stessa necessità di rispetto della legge di bilancio, e

eppure verranno spesi per oltre 4 miliardi di euro ancor prima che la legge di assestamento sia votata. C'è una continua violazione della legge di contabilità.

Il senatore Baldassarri ha citato Vittorio Emanuele Orlando ed io, a questo punto, citerò Bartali, visto che il Presidente del Consiglio continua a definirsi, in modo insistente e sedicente, un cultore del ciclismo.

Tutti i congressisti gli dissero di darsi all'ippica. A questo punto, se non si vuole dare al ciclismo, che il Governo si dia all'ippica.

la normativa che presidia l'emanazione dei decreti-legge e l'attenzione che tutti gli organi che contribuiscono alla nascita e al percorso di un provvedimento del genere dovrebbero porre in materia. Questo decreto-legge sicuramente è assolutamente disomogeneo. Inviterei, pertanto, i colleghi, soprattutto quelli di maggioranza, a dare una scorsa ai titoli degli articoli che compongono il decreto-legge, che è stato arricchito

proroga un'altra già esistente in finanziaria, la quale viene - appunto - sostituita dall'articolo 16, e che pertanto l'urgenza riposa nello stesso concetto di proroga di un termine peraltro già scaduto. Voglio far presente all'Assemblea (anche perché resti agli atti la mia obiezione che rappresenta un ulteriore motivo di contestazione con efficacia di pregiudizialità

vengano delegificate, cioè si trasformino in norme regolamentari che il Governo dovrà adottare con provvedimenti successivi. Confermo,

il Parlamento in qualche modo delega, attraverso la redazione di un regolamento di delegificazione, il Governo ad approvare norme che sostituiscono norme di legge entro il termine

e specifica motivazione. Ho apprezzato l'espressione del collega Baldassarri che ha definito questo decreto-legge un delitto finanziario. La mia anzianità d'Aula mi consente di ricordare

un'opinione legittima, ma che la maggioranza non condivide. Poi si può discutere, da un punto di vista puramente dottrinario, su quale possa essere l'incidenza eventuale di un contrasto di una norma di legge successiva

nel senso dell'accoglimento di una pregiudiziale che interromperebbe - com'è ovvio - l'*iter* di formazione di quest'atto. Gli argomenti, invece, che pongono tecnicamente una pregiudiziale di costituzionalità sono quelli

Alle due questioni sottolineate dal collega Pastore credo che si possa rispondere nel seguente modo: siamo di fronte ad un atto che, sostanzialmente, è una piccola manovra di finanza pubblica; è chiaro che attiene - com'è stato ricordato - all'utilizzazione delle risorse che si sono rese disponibili. È del tutto ovvio che un atto che si pone questo fine, intrinsecamente, ha una molteplicità di obiettivi da raggiungere. In questo caso, la disomogeneità, che è sicuramente un elemento di rilievo dal nostro punto di vista, non può essere data semplicemente dalla lettura dei titoli degli articoli articoli che, inevitabilmente, avranno oggetto diverso e molteplice, ma dovrà essere ritrovata nel fine complessivo dell'atto nel quale ciascun segmento si inserisce.

Questo vuol dire che non basta capire che c'è un lasso di tempo prima che il regolamento si adotti; la legge oggi stabilisce che il regolamento può essere

possibile fare, ecco che il ragionamento del collega Pastore non è idoneo a sostenere l'argomento dell'incostituzionalità. Per tali motivi, signor Presidente, raccomando all'Aula di respingere le questioni pregiudiziali.

poche parole per replicare alle spiegazioni che i colleghi senatori dell'opposizione hanno voluto offrire a quest'Aula per argomentare le questioni che hanno posto in termini di pregiudizialità sia di carattere procedurale, sia di carattere costituzionale. Gli argomenti che vengono offerti sono tutti interessanti, alcuni suggestivi, alcuni meritano una replica puntuale. Ho annotato le osservazioni dei colleghi Baldassarri e Ferrara e convengo con quanto ha detto il collega Villone, che molte delle questioni poste,

se una norma possa modificare, rispetto ad una norma precedente della legge finanziaria, i princìpi e le regole della contabilità dello Stato. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia deformazione professionale, più volta agli aspetti istituzionali che a quelli finanziari, mi impone una replica solo sotto questo profilo: l'articolo 77, comma primo, della Costituzione precisa che il Governo è delegato ad emanare decreti-legge aventi valore di legge ordinaria. ordinaria. Questo basterebbe per dire che non si può porre alcuna questione con riferimento a leggi che hanno un'eguale forza vincolante che vengono emanate successivamente; quindi tale argomento, quantunque suggestivo, e cioè se vi debbano essere leggi ordinarie che abbiano una forza cogente maggiore rispetto alle altre, può essere facilmente confutato alla luce di questa semplicissima argomentazione che fa riferimento all'articolo 77, comma primo. Ciò non significa che le questioni che vengono poste non siano rilevanti, tuttavia il riferimento che c'è in una legge ordinaria al DPEF, quanto ai vincoli di contabilità, è una scelta che può essere discussa, può essere ritenuta nel merito inappropriata, si può ritenere in deroga ad altre leggi dello Stato, ma dal punto di vista della pregiudizialità, a mio avviso, non esiste un fondamento. Gli argomenti che invece presta all'Aula il senatore Pastore hanno una maggiore pregnanza sotto il profilo delle questioni di costituzionalità; per i profili di disomogeneità del testo vale l'argomento del collega Villone: non possiamo guardare i titoli,

che è apparentemente una norma di non immediata efficacia, perché rinvia ad un regolamento da adottare entro il 30 ottobre 2007. La sequenza delle leggi nel tempo ed il riferimento al comma 989 della legge finanziaria, tuttavia, ci chiariscono che si tratta della proroga di un termine già scaduto 90 giorni dopo l'entrata in vigore della finanziaria, che quindi riapre

ovvero l'idoneità dello strumento di delegificazione. Signor Presidente, l'articolo 17, comma 2, prevede che non già il Ministro, ma il Governo possa emanare regolamenti di delegificazione nell'ambito di quella che è la struttura dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Ciò è possibile, come diceva il collega Villone, solo nell'ambito di una legge emanata dallo Stato che conferisca al Governo questa possibilità. il collega Pastore c'è una sostanziale innovazione rispetto al comma 989 della legge finanziaria. Voglio ricordare che stiamo parlando di tasse e tributi e che l'articolo 23 della Costituzione, che forse avrebbe dovuto essere appropriatamente citato in quest'Aula, prevede una riserva relativa, e non assoluta, di legge. Tant'è che è consentito che tasse e tributi vengano messi anche a livello regionale e a livello locale. Questa riserva relativa di legge - dice sempre la Costituzione - ha bisogno che venga esercitata nell'ambito di una discrezionalità tecnica. E perché questa discrezionalità tecnica sia correttamente esercitata è necessario che la legge preveda dei criteri e dei riferimenti ai princìpi direttivi emanati dalla legge stessa. Questa è la ragione unica

che non vi sia alcun problema in termini di pregiudizialità di carattere procedimentale, per le ragioni di merito che ho detto, e che non vi sia alcuna pregiudizialità di carattere costituzionale che possa essere opposta rispetto a questo provvedimento. È per questo

Presidente, in questi giorni si parla tanto di test. Se si potesse fare un test di onestà

Mi sembra che gli uffici abbiano fatto un ragionamento lineare, molto trasparente ed onesto. Ricordava il Presidente che per la prima volta credo che informalmente la collaborazione ci sia sempre stata, e di questo li ringraziamo - gli uffici hanno fatto degli appunti puntuali. al primo, come già ricordato, stiamo facendo riferimento, come copertura, ad un documento di assestamento che deve arrivare. arrivare. Si dice che la madre sia certa e che il padre, di solito, sia incerto. Qui abbiamo una madre sicura, la spesa,

va sempre a prendere nelle tasche dei soliti contribuenti che, caso strano, di solito risiedono al Nord, vi dico che siamo stufi di avere un metro che vale per il Governo e per lo Stato che prevede

per forza, con gli accertamenti preventivi, dichiarare e garantire che, a prescindere, hanno guadagnato una determinata cifra, altrimenti vengono loro mandati gli sgherri di Stato che troveranno sicuramente qualcosa che non va, concludendo con il patteggiamento.

i contribuenti del Nord non riscuotono neanche l'attenzione di qualcuno della maggioranza. Quando poi però dovete presentare il Partito Democratico o raccontare delle fole venite a Torino e al Nord. Ma state tranquilli

un'entrata certa e tirando i parametri di elasticità, come volete voi. Questo non è un Paese serio. Questo è il Paese delle banane. Per questo, Presidente, auspichiamo con forza l'accoglimento delle questioni pregiudiziali e le chiediamo di rimandare in Commissione il provvedimento.

ossia quelle norme con forza di legge che possono essere poste con le stesse modalità delle leggi ordinarie ma non possono essere derogate. Tra le fonti atipiche vi è la legge di contabilità che, tra l'altro, richiama direttamente l'articolo 81 della Costituzione, essendone attuativa. Basta leggere l'articolo 11-*ter*, dove si dice che, in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il sistema delle coperture dei provvedimenti di spesa è tipizzato e non può essere derogato da leggi ordinarie. Poiché il decreto-legge che stiamo esaminando all'articolo 1 deroga proprio all'articolo 11-*ter* della legge di contabilità, cioè al sistema delle coperture delle leggi ordinarie, in questo caso si pone in contrasto con la Costituzione. Questo decreto-legge è sostanzialmente scoperto, motivo per il quale siamo favorevoli alla questione pregiudiziale, ritenendosi che in ogni caso il Parlamento non debba approvare una legge scoperta anche se l'ha approvata il Governo ed anche se - mi domando come - il Presidente della Repubblica ne ha autorizzato la presentazione alle Camere. Per tali motivi, siamo favorevoli alle questioni pregiudiziali presentate.

Presidente, questa mattina non abbiamo avuto in Aula un relatore al provvedimento e la discussione è iniziata con un'introduzione del Presidente della Commissione bilancio. È una situazione eccezionale e straordinaria perché normalmente per ogni provvedimento vi dovrebbe essere un relatore.

che nella Commissione bilancio il provvedimento non è stato esaminato per intero e non si è potuto completare l'esame degli emendamenti.

il nostro Regolamento non contempla tale possibilità. La Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito che un dato argomento doveva essere discusso un determinato giorno

ho capito.

**Il Senato non approva.** Chiariamoci bene. Io su questo discorso del chiudere o meno, dinanzi alle urla che si sentono in Aula, invito i senatori - perché sempre di questo si tratta - a controllare perché a questo mi riferisco. Infatti, rispetto alle vostre segnalazioni, c'era una scheda cui non e ho provveduto a farla togliere. Se urliamo, non si capisce nemmeno la richiesta che legittimamente un senatore può fare. Non è questione di tempi della durata della votazione. FERRARA

Se durante la votazione l'Aula offre lo spettacolo di oggi, nessun Presidente è in grado di capire l'obiezione che viene rivolta. *(Commenti

il senatore Ferrara farebbe bene a dare un'occhiata ai banchi della sua parte perché purtroppo anche per questo voto e per l'ennesima volta vi sono senatori che votano a doppio, a triplo e a quadruplo e questo non va bene.

a indicare il punto dove intervenire? Questo riguarda tutta l'Aula. Il silenzio è una condizione essenziale per poter intervenire. È chiaro il discorso? Noi metteremo - spero - immediatamente durante le ferie i posti fissi

sono un senatore quieto, ma osservatore: credo che

Qualche mese fa, durante una di queste gazzarre, una scolaresca stava assistendo alla seduta: mi sono vergognato di essere senatore della Repubblica.

in confronto al discredito che questo tipo di votazioni getta su di noi. Il voto digitale si può fare: non si può lasciare il dito in Aula, che non può votare da solo, non può essere prestato ad un collega né può essere usato da un altro

Presidente, qualcuno ha definito gazzarra quanto è accaduto pochi minuti fa, in occasione del voto.

legittimo rappresentante, costano allo Stato 258,23 euro. Bisognerebbe che venissero ritirate quando il senatore è assente e sono inserite senza la sua presenza.

Abbiamo osservato ieri sera al senatore Boccia che il pregiudizio a che ciò avvenga non è tanto costituito da un' azione dilatoria, ma dal fatto che il Governo si è prodotto negli ultimi tempi in una richiesta, o in una prevista richiesta, di fiducia sui provvedimenti in esame. Ciò lascia poco spazio all'opposizione, perché è chiaro che l'interesse dell'opposizione potrebbe essere anche quello di avere un relatore

l'opposizione si trova nella necessità di non adire a tale richiesta e quindi questo finisce per essere un evento corrosivo del normale *iter*, di cui ci di cui ci dispiacciamo, ma non crediamo che le pregiudiziali di ragionamento e la richiesta di modifica del Regolamento possano essere poste tra le ipotesi di cui alla richiesta fatta dal senatore

*(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a trattare gli argomenti connessi al mio ordinario lavoro di Commissione, dato che il decreto oggi al nostro esame contiene anche alcune misure relative all'agricoltura e alla pesca: confesso che la cosa mi meraviglia un po', considerato che il Governo Prodi ci ha abituati al suo cronico disinteresse per il secondo settore della nostra economia. Quando il Governo si è accostato al settore, gli effetti hanno destato viva preoccupazione presso gli addetti, quando non lo sconforto e la protesta. Leggendo più attentamente il provvedimento, mi accorgo che alcune misure costituiscono atti dovuti, senza l'adozione dei quali si rischierebbe di esasperare ulteriormente la situazione critica in cui si trovano ad operare le imprese agricole, della pesca e dell'acquicoltura. Altre misure, invece, cercano di tamponare emergenze create in vari casi dal Governo con scelte politiche sbagliate e con misure di attuazione oltre il limite dell'aberrazione. Devo per altro sottolineare che il passaggio alla Camera ha consentito, per certi versi, di modificare in senso migliorativo il contenuto del decreto. Ed è proprio con l'intenzione di contribuire a migliorare ulteriormente il provvedimento che abbiamo presentato alcuni emendamenti all'articolato riguardanti la pesca e l'agricoltura. Il nostro intento sarà ovviamente frustrato dall'annunciato ennesimo voto di fiducia: del resto, il Governo ha ormai perso la fiducia del Paese e quindi ricorre sempre di più al voto di fiducia in Parlamento Volendo esaminare alcune delle disposizioni recate dall'articolo 15, osserviamo che la dotazione annuale del fermo biologico dell'attività di pesca prevista al comma 1 rappresenta un atto dovuto finalizzato ad assicurare il sostegno per i marittimi imbarcati con effetto di ammortizzatore sociale. Quindi nulla di particolarmente innovativo rispetto al passato; non vedo un minimo tentativo di procedere lungo l'auspicata direzione di garantire una pesca sostenibile dal punto di vista sociale ed economico, oltre che ambientale. In questo caso, i tanti Soloni dell'ambientalismo marino nostrano sono rimasti muti come pesci, mentre ricordo che durante gli anni del nostro Governo questa era la stagione in cui essi si scatenavano in previsioni apocalittiche sulla persistenza degli *stock* ittici. Per quanto concerne invece le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 che rinviano fino al 30 novembre 2007 la scadenza per il completamento delle operazioni di autotutela o di presentazione dei ricorsi alle commissioni tributarie al fine di correggere errori sulle variazioni catastali, qui siamo in presenza del più caratteristico degli esempi di una norma attesa ed ormai indispensabile ed indifferibile, che tuttavia pone soltanto temporaneo rimedio ai problemi creati in questo contesto dal Governo Prodi. Ricordiamo, infatti, e lo facciamo con autentico disgusto, che l'operazione di aggiornamento delle rendite catastali è stata impostata con efficacia retroattiva e tenendo conto solo delle variazioni in aumento, e non in diminuzione, ovviamente, degli estimi, con il risultato, ormai pratica consueta per questo Governo delle tasse, di sovvertire i più elementari princìpi del corretto rapporto tra amministrazione fiscale e contribuente. Occorre ricordare che il settore agricolo italiano soffre di cronica sottocapitalizzazione, che i redditi agricoli sono in costante decremento, che i costi di produzione continuano a crescere anche perché in parte legati al prezzo del petrolio, che la concorrenza internazionale - anche quella intracomunitaria - è pressante, che la riforma della politica agricola comunitaria recentemente introdotta determina ulteriore riduzione dei margini di contribuzione; occorrerebbe ricordare tutto ciò, prima di aumentare le tasse degli agricoltori, ma - per contro - il Governo attuale ha proceduto in modo penalizzante. E lo ha fatto per un anno intero, contraddicendo sé stesso molte volte, tassando anche il capitale fondiario, il mezzo produttivo imprescindibile, cioè la terra. Come dimenticare le tutt'altro che profetiche dichiarazioni del buon De Castro il quale, solo pochi mesi fa, si impegnava ufficialmente per l'invarianza fiscale per l'agricoltura? E lo scriveva, e lo diceva ripetutamente in Commissione, e lo proclamava addirittura nei convegni organizzati da partiti di Governo. Ricordo anche che, in occasione di uno di questi convegni (quello organizzato dall'Udeur), lo sfidai a dimostrare di contare, lui Ministro, un po' di più di un Vice Ministro con delega al fisco. Ho vinto la scommessa, ma posso assicurarvi che avrei preferito perderla! Qui siamo invece oltre il patetico: si tenta maldestramente di infinocchiare gli agricoltori e di far passare come un beneficio per il settore quello che altro non è che la correzione in corsa degli effetti di questa sconsiderata operazione fondata, tra l'altro, sul ricorso ad una discutibilissima procedura automatizzata che è risultata viziata da errori macroscopici compiuti dall'Agenzia del territorio, Agenzia che naturalmente dipende da Visco. Si tratta di errori tali da determinare in molti casi assurdi ed ingiustificabili cambiamenti addirittura delle qualità catastali, con conseguenze insostenibili per gli agricoltori in termini di inasprimento degli estimi. Vogliamo parlare delle coltivazioni di pomodoro da industria diventate, come per incanto, orti irrigui, oppure delle coltivazioni a secco di soia e mais diventati seminativi irrigui? Sono miracoli di Visco anche questi. In tali casi si fatica a distinguere la volontà persecutoria dall'ignoranza e dalla stupidità: spesso però le due caratteristiche non si escludono a vicenda, bensì si potenziano. Accogliamo invece con favore la modifica apportata dalla Camera dei deputati con l'inserimento del comma 1-*bis*, che stabilisce l'estensione al settore della pesca del credito di imposta, rimediando ad una lacuna dell'ultima finanziaria che aveva escluso proprio questo settore da tale beneficio. Per il resto, ci troviamo di fronte alle proroghe di norme dilatorie come nel caso dei termini per la ricognizione della situazione debitoria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia: non mi pare nulla di trascendentale. Per quanto concerne le nostre proposte emendative, voglio ricordare che il settore della pesca è da tempo in attesa dell'introduzione sperimentale del regime IVA speciale che il Governo Berlusconi aveva varato, agevolazione di perequazione con l'agricoltura che purtroppo è stata abbandonata senza essere stata attuata, né più riproposta dal Governo. E non ci si venga oggi a raccontare che non è pervenuta l'autorizzazione di Bruxelles (anzi, ci è già stato raccontato da De Castro più volte) e che dunque si incorrerebbe nella mannaia di una procedura d'infrazione. Ricordo, per esperienza personale, che quando assunsi l'onere di governare la pesca italiana ereditai ben cinque procedure d'infrazione dai Governi della sinistra, che abbiamo felicemente risolto una dopo l'altra. Basta avere un minimo di volontà, un minimo di perseveranza, rapporti di collaborazione autentici e non solo dichiarati con le autorità comunitarie e una decorosa capacità di muoversi in Consiglio dei ministri europei: tutte caratteristiche che vedo penosamente mancare all'odierno Esecutivo, ancorché presieduto da un *ex* Presidente di Commissione dell'Unione Europea. Temo che in realtà il Governo non intenda proprio mantenere questa promessa ai pescatori professionali e dunque si avventuri in spiegazioni puerili che però suonano come ligio ossequio alle norme comunitarie. Spero che i pescatori non si facciano imbrogliare e pretendano, attraverso le loro associazioni, che De Castro provi ad assumere un comportamento meno incline al cedimento. Ricordo di aver inventato l'equiparazione tra pescatori ed agricoltori in materia di IVA, ricordo di aver passato le notti a Bruxelles per difendere il reddito e l'esistenza stessa dei nostri pescatori - credo di non aver fatto nulla di eroico ma di doveroso - ed ora è veramente deprimente vedere la delegazione italiana così prona ai *diktat* degli eurocrati: uno spettacolo realmente deplorevole. Perciò, abbiamo proposto una modifica legislativa che renderebbe direttamente applicabile la norma auspicata. Il comparto ittico ha necessità urgente di ulteriori misure di sostegno. Abbiamo proposto la sospensione dell'applicazione degli studi di settore, abbiamo proposto altri esempi di semplificazione come l'istituzione di sportelli unici, abbiamo proposto tutta una serie di misure, signor Presidente, che evidentemente

che questo Esecutivo, ormai sfilacciato e degradato al livello di *ring* tra pugili suonati che si lanciano gli stracci, sia nelle condizioni di accogliere ciò che a noi pare francamente ragionevole e dubito anche che abbia la sensibilità politica o la lucidità di accorgersi che il mondo agricolo e della pesca è arrivato ben oltre il limite della sopportazione: nei prossimi mesi vedremo gli effetti di questo immobilismo tragico ed infingardo.

l'ipotesi di riduzione del debito votata nel DPEF dello scorso anno e concordata con l'Unione Europea: infatti, si chiude al 2,5 per cento invece del 2,8 per cento Tutto ciò è stato reso possibile sia in relazione ad una situazione più favorevole dell'economia, sia soprattutto al favorevole andamento delle entrate fiscali dovuto in particolare alla lotta all'evasione. Anche qui - lo voglio dire con pacatezza

sicuramente ha pesato positivamente un indirizzo che fin dai primi provvedimenti del luglio scorso fu dato da questo Governo e da questa maggioranza, ma soprattutto dall'idea forte non ci sarebbero stati più condoni e quindi ognuno si è dovuto adeguare a questo nuovo clima. È una scelta politica chiara - lo vorrei ripetere - e rigorosa quella fatta dal Governo,

che avrebbero preferito destinare tutto l'extragettito alla riduzione del debito, senza capire che questa scelta rende possibile un aumento delle pensioni minime (900 milioni nel 2007, 1.500 nel 2008 e nel insieme ad altri interventi sociali di cui, per brevità, ne ricordo solo alcuni: il fondo globale per la lotta all'AIDS che ci vedeva inadempienti come Paese in tutti gli organismi internazionali, misure rivolte ai giovani come il riscatto della laurea e la congiunzione dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali, tutte misure che si configurano

del tutto evidente che questi seppur limitati aumenti delle pensioni minime si tradurranno tutti - ripeto, tutti - in aumento dei consumi e conseguentemente anche delle entrate per lo Stato. Non mi soffermo sugli aspetti riguardanti gli enti locali, in particolare sull'attenuazione del Patto di stabilità per poter utilizzare gli avanzi, o sui provvedimenti riguardanti la scuola e l'università, o ancora - nessuno lo ha ricordato - sull'impegno mantenuto di trovare una copertura

Ebbene, ritengo che questa applicazione sia stata sia formale che sostanziale, in primo luogo perché la natura della misura sulle pensioni ha un carattere di miglioramento delle condizioni per i soggetti appartenenti alle fasce sociali più deboli, e quindi anche indirettamente diminuisce la pressione fiscale; in secondo luogo perché rende ancora più evidente una scelta politica,

Quando si coniuga rigore con equità e sviluppo la coalizione è più unita, così come la maggioranza dell'Unione. Si applica il programma; si poteva - a nostro avviso - avere più coraggio anche lo scorso anno spalmando in due anni la manovra

perché con recepimento integrale di una mozione votata in quest'Aula - ecco il contributo del Senato a questa normativa che stiamo, spero, per approvare - diventa norma l'ordine del giorno sugli indicatori di normalità costruito in Commissione finanze in Senato, approvato da quest'Aula; da considerarsi indicatori sperimentali e senza nessun automatismo accertativo. meglio il collega Bonadonna, ma vorrei sintetizzare come segue: si è passati da quel patto scellerato con queste categorie del ceto medio e delle professioni degli anni '60, che in qualche modo scambiava consenso, ad un certo tipo di sistema di potere con evasione fiscale tollerata; oggi invece si può lavorare a un nuovo patto che in qualche modo la mozione

positivi che lo compongono lo rendono importante e - come ho già detto - fortemente intrecciato alla manovra economica che preparerà una finanziaria di crescita e di sviluppo, e noi speriamo e lavoriamo perché sia tale. Ma voteremo a favore anche perché - mi sia consentito di concludere con una battuta vogliamo ricordare che ogni procedura di ravvedimento operoso ha sempre un termine, superato il quale in assenza di una soluzione positiva si iniziano procedure di tipo conflittuali.

qualche tema di particolare interesse ed addirittura qualche tema curioso. È il caso del comma 7 dell'articolo 6, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo speciale per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone confinanti tra le Regioni. Questa è la motivazione ufficiale, ma la vera intenzione del Governo emerge se si valuta la portata finanziaria del provvedimento: si tratta di 20 complessivi, di cui 14 milioni destinati - questo è il lato interessante - ai Comuni appartenenti a Regioni a statuto ordinario confinanti con Regioni a statuto speciale. Rientrare nelle zone elette non è facile: occorre ottenere un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'appoggio del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Questo provvedimento, apparentemente generico, ha un nome e un cognome per chi lo sa leggere. Io provengo dal Trentino e lo leggo nel seguente modo: la diaspora minacciata da alcuni Comuni del Veneto, attirati da considerati e sedicenti *Eldorados* del Trentino e dell'Alto Adige, ha sicuramente ispirato questa iniziativa del Governo che corre, quindi, ai ripari per salvare confini che sono difesi dalla Costituzione e per scongiurare altri *referendum*, dopo quelli che si sono già effettuati e che hanno sancito da parte degli abitanti del Veneto una preferenza schiacciante bulgara per il passaggio al Trentino. C'è la convinzione che gli statuti delle autonomie speciali, sia regionali che provinciali, consentano una migliore distribuzione delle risorse e soprattutto dispongano di più risorse da distribuire rispetto alle Regioni a statuto ordinario. In realtà, 14 milioni di euro su 20 milioni di euro complessivi non sono un granché, se si pensa alla vastità dei territori che confinano con le tre Regioni a statuto speciale in terraferma, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (ipotizzando che, per quanto riguarda le due Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, non vi siano confinanti che rivendicano qualcosa). Il movente di questi tentativi di fuga da una Regione ordinaria ad una a statuto speciale non è soltanto la ricerca di un pacchetto più cospicuo di risorse; spesso il dissenso di partenza deriva, magari per la perifericità geografica di queste zone, dalla scarsa considerazione in cui sono tenute da parte delle Regioni di appartenenza. Chiaramente la protesta viene alimentata dalla vita quotidiana e, quindi, dal confronto con i vicini che stanno appena al di là dei confini, che evidentemente ostentano maggiori disponibilità con interventi sia pubblici che per le iniziative private. Proprio oggi è apparsa su un giornale del Trentino la notizia

si dimostra che in effetti i soldi sono talmente tanti che ci si può permettere addirittura di darli ai vicini di casa, peraltro senza alcuna protesta dei legittimi proprietari e titolari di questi denari che sono i trentini.

Signor Presidente, intendo utilizzare i pochi minuti a mia disposizione per recuperare il senso di una critica che noi di Forza Italia, dall'inizio di questa legislatura, formuliamo nei confronti della politica economico‑finanziaria del Governo Prodi. Una critica che è finalizzata a dimostrare che il Governo, nei dodici mesi di attività, a parer nostro, non solo non ha risolto, ma neppure affrontato, i problemi veri dell'economia del nostro Paese. Ricordo per sommi capi, signor Presidente, alcuni passaggi che ritengo importanti, al fine di dimostrare il senso di questa critica. Appena insediato il Governo Prodi, il Governo Prodi, il ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa lanciò l'allarme sui conti pubblici, arrivando financo a dire che la finanza del nostro Paese era tornata all'inizio degli anni Faccio presente che nel 1992 - allora sì - si toccò il baratro a livello di conti pubblici del nostro Paese. Ovviamente, nei mesi successivi, si è capito che tutto questo non era vero, non era vero, anche se, nel secondo appuntamento, il ministro dell'economia Padoa-Schioppa, presentando il Documento di programmazione economico-finanziaria, promise che si sarebbe intervenuti sulla spesa strutturale del nostro Paese aggredendo il tema delle pensioni, della sanità, del pubblico impiego e degli enti locali. Si è visto poi, in sede di finanziaria, che nessuna delle riforme proposte ha trovato un'iniziativa da parte del Governo. Successivamente, il Governo si è impegnato nella discussione in Parlamento del cosiddetto decreto Bersani-Visco, presentato - per la verità - con molta enfasi, in ordine alle questioni sulle liberalizzazioni volute da Bersani sui taxisti, i farmacisti e i notai (poi si è visto come siano andate le cose) e cercando in tutti i modi di passare sotto silenzio le norme antievasione di Visco, quelle sì, a nostro Poi il Governo ha presentato la legge finanziaria per il 2007. Purtroppo, in coerenza con l'impostazione cara alla sinistra e, ovviamente, in contraddizione con le denunce del ministro Padoa-Schioppa fatte all'inizio della legislatura, nessun taglio alla spesa pubblica è stato ordinato e nessuna riforma strutturale è stata avviata: si è trattato soltanto di approvare e proporre al Parlamento un aumento generalizzato della pressione fiscale, non solo a carico dei precettori dei redditi medio-alti, ma di tutti.

È la via percorsa negli anni Novanta, quando si tentò il riequilibrio dei conti pubblici attraverso l'inasprimento della pressione fiscale, con il risultato che si è aggravata la situazione dell'economia italiana nel suo complesso rispetto ad altri Paesi più

finanziaria dello scorso anno, unitamente a due fattori tra di loro interconnessi, ha reso ancora più problematica la situazione del nostro apparato produttivo. Tali fattori sono la minore solidità della nostra struttura produttiva, a confronto con Germania, Inghilterra e Francia, e un apparato produttivo sempre più frammentato per la presenza consistente delle piccole e medie imprese. Non ci stancheremo di dire, signor Presidente, che l'economia nella lira era una cosa, ma l'economia nell'euro postula comportamenti alternativi, perché in essa sono i fattori reali della produzione che stabiliscono la competitività di un sistema, e quindi di un sistema produttivo. Nell'economia della lira, lo ricordiamo, c'erano le svalutazioni competitive che ci aiutavano e ci hanno consentito allora di trasformarci da Paese prevalentemente agricolo in un Paese industriale assai evoluto. In queste condizioni, l'economia italiana, a partire dagli anni '90, non è riuscita a trarre beneficio dalla forte espansione del commercio internazionale, proprio a causa della rilevante perdita di competitività

la finanziaria del 2007 e la politica di bilancio che ne è conseguita fino ad oggi e che viene riproposta nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nel provvedimento oggi in discussione, perché ritenevamo non adeguata all'esigenza della politica la scelta di seguire un rigore fine a sé stesso, cioè una riduzione di disavanzo al di sotto del 3 per cento conseguita solo e soltanto aumentando delle entrate. signor Presidente, non si è inciso sulle cause che sono all'origine della bassa crescita dell'economia italiana, perché è vero che nell'area dell'euro si sta registrando una sensibile ripresa, ma non sfugge a nessuno che la ripresa registrata in Italia è assai inferiore rispetto a quella che si registra in Germania, in Francia, in Inghilterra e in Spagna. Per questo siamo stati critici, come siamo stati critici sul Documento di programmazione economico-finanziaria, perché per noi è una scommessa sulla crescita che è tutta da dimostrare. Mancano i presupposti per credere in una crescita vera e reale del nostro apparato produttivo. riferito alla riforma dei servizi pubblici locali che è su un binario morto, non parlo della liberalizzazione dell'energia che ancora deve diventare legge; concludo facendo alcune puntuali osservazioni sul provvedimento oggi al nostro esame, il famoso tesoretto. Per noi è semplice costruire una critica: ci attestiamo alle osservazioni puntuali e precise che ha fatto il governatore della Banca d'Italia Draghi e che hanno fatto i centri di studio e di ricerca più avanzati d'Europa e del mondo. Dice il governatore Draghi: «Con il debito pubblico che abbiamo, con un disavanzo strutturale pari al 3 per cento del PIL, con gli oneri previdenziali certi, impliciti all'andamento della demografia del nostro Paese, non esiste un tesoretto da spendere». È un'illusione ottica, quella che ci propone il Governo con questo provvedimento. in parte al miglioramento del ciclo economico inferiore a quello degli altri Paesi e in parte al parziale successo dell'azione di recupero della base imponibile, oggi le condizioni suggerirebbero, signor Presidente, di parlare e di operare per una riduzione delle imposte, perché c'è un problema di competitività fiscale con gli altri Paesi d'Europa, e soprattutto c'è un problema che in termini più robusti andrebbe affrontato, che è quello di aiutare davvero le imprese a recuperare competitività. In qualche modo, avreste dovuto seguire l'esempio tedesco, come ormai tutti sanno, l'esempio di un Paese che ha contenuto la spesa pubblica, che ha ridotto il rapporto tra spesa pubblica e PIL senza pregiudicare la spesa sociale, un traguardo che secondo noi era ed è a nostra disposizione, bastava avere la volontà politica e non farsi condizionare dalla consorteria del partito della spesa pubblica che, come ben sappiamo, si annida nei partiti di sinistra, nei sindacati, nei mille rivoli nei quali viene viene organizzata la spesa pubblica nel nostro Paese. Per questo noi non possiamo che essere contrari alle norme proposte con il decreto in discussione quest'oggi e siamo in buona compagnia nell'esercitare questa critica, perché riconosciamo validità alle osservazioni della Banca d'Italia, alle critiche del Fondo monetario, alle opinioni critiche della Commissione dell'Unione europea, ai rilievi critici dell'EUROSTAT e dell'ISAE, di centri qualificati che hanno stigmatizzato questa scelta assolutamente demagogica che non serve all'economia del Paese e soprattutto non è funzionale ad una politica di sviluppo e di crescita. Di fronte a spese correnti in crescita, ad una pressione fiscale sempre sostenuta e ad un debito pubblico che non accenna a diminuire, il vantaggio che ci dava l'extragettito avrebbe dovuto essere utilizzato

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo decreto-legge suscita molte perplessità, sia di ordine politico che di ordine tecnico. Si tratta sicuramente di una normativa manifesto, volta a soddisfare le esigenze politiche della sinistra comunista che, dopo la fallita manifestazione di protesta a Roma, ha voluto recuperare un rapporto con la propria base elettorale a spese dello Stato. Questo provvedimento infatti non ha i requisiti dell'urgenza e della necessità, è *omnibus* ed è infondato dal punto di vista costituzionale, perché viola palesemente l'articolo 81 della Costituzione, come pure abbiamo visto ieri. Prima questione: i 16 articoli mirano ad utilizzare, con una misura di spesa, pari a 4 miliardi e 700 milioni dei dei 7 miliardi 403 milioni di euro di maggior gettito tributario, rispetto alle previsioni fatte al 31 dicembre 2006, ossia rispetto alla relazione previsionale programmatica. La vicenda aperta è che i 7 miliardi e mezzo di euro non sono ancora stati registrati nel bilancio dello Stato, perché l'assestamento di bilancio non è stato ancora approvato. Chiunque abbia un minimo di conoscenza delle fondamentali regole di contabilità, sa che non possono essere spese risorse che non sono iscritte a bilancio. Sicché, con l'uso del tesoretto, attraverso un decreto-legge, quindi immediatamente efficace, applicativo della normativa in questione, si spendono somme non risultanti disponibili nel bilancio dello stato. L'urgenza politica è prevalsa sul rispetto della legge e del diritto costituzionale. Non mi sembra una buona pratica politica. Seconda questione: si usa il termine tesoretto per indicare una somma, 4 miliardi e 100 milioni di euro, come dicevo, quale sopravvenienza attiva rispetto ad una previsione che non è stata enumerata tra le entrate tributarie. Si tratta in realtà di un saldo netto positivo nel bilancio dello Stato? Assolutamente no! Con la legge finanziaria del 2007 è stato modificato il bilancio sul lato della spesa attraverso un incremento di risorse, in parte finanziate con nuove e maggiori entrate, in parte attraverso l'indebitamento, cioè chiedendo prestiti sui mercati finanziari. Sicché, se dopo sei mesi ci si è accorti che le entrate erano maggiori di quelle previste, sarebbe stata buona politica utilizzarle per ridurre il debito contratto con la stessa finanziaria 2007. Invece di tutto questo, il maggior gettito tributario si usa per ulteriori spese, pari appunto a 7 miliardi e 403 milioni di euro,

Terza questione: le spese previste dal decreto-legge in esame sono strutturali, cioè ripetibili nel tempo, mentre l'extragettito di cui si parla è stato registrato nell'anno in corso. Quanta parte di entrate tributarie è strutturale, ossia ripetibile nel tempo, per finanziare una spesa che è ripetitiva? Lo abbiamo chiesto in più sedi e a viva voce, ma nessuno della maggioranza e del Governo ha saputo dirci quanta parte dei 7 miliardi e 403 milioni di euro è entrata strutturale e quanta dovuta alla componente ciclica, ossia alle favorevoli condizioni di crescita del PIL, che quest'anno si attesta al 2 per cento, ma che nel 2008 è stimato all'1,7 per cento? In tal senso non sono state convincenti alcune argomentazioni dell'onorevole Visco in Commissione qualche giorno fa. Accanto a queste considerazioni c'è inoltre un *refrain* che la maggioranza porta avanti in tutti i discorsi: si tratta di recupero di evasione fiscale! Quindi è entrata strutturale. Se è vero quello che ha sempre sostenuto ogni Ministro dell'economia e delle finanze, che, posto 100 il valore di un accertamento fiscale, lo Stato dopo alcuni anni riesce ad incassare 10 di questo 100, come è possibile ipotizzare un risultato così repentino in appena dodici mesi di Governo e appena otto mesi dai provvedimenti fiscali antielusivi? concesso il miracolo di Visco, come giustificano nel contempo i colleghi del centro-sinistra l'aumento di mezzo punto, cioè dal 42,3 al 42,8 per cento, della pressione fiscale per il 2008 Se le maggiori entrate sono da recupero di evasione fiscale, ossia dall'allargamento della platea dei contribuenti, non ci dovrebbe essere aumento di pressione fiscale, ossia l'aumento delle tasse per chi già le paga. Si tratta, a ben vedere, di propaganda politica: il Governo Prodi è il Governo delle tasse e della spesa allegra. Basti vedere l'articolo 7 del decreto-legge n. 81, laddove si autorizzano ben 2 miliardi di euro di spesa per coprire capitoli di spesa che erano stati ibernati (i famosi accantonamenti disaccantonati) come forma surrettizia di tagli in quanto avrebbero dovuto generare, a fine anno, economie pari a 4 miliardi e 100 milioni di euro per allentare il disavanzo dello Stato. Secondo il comma 507 della legge finanziaria 2007, queste economie si sarebbero ottenute attraverso una riqualificazione della spesa, ossia eliminando la spesa inutile ed improduttiva, ovvero spendendo meglio gli stanziamenti esistenti, proprio come dite voi del centro-sinistra. Dopo appena sei mesi, vi siete accorti che al massimo avreste potuto risparmiare, di quei 4 miliardi e 100 milioni, soltanto 2 miliardi e 100 milioni e avete pertanto rifinanziato per 2 miliardi la spesa. Se è vero questo fallimento sulla vostra capacità di risparmiare, come potete essere credibili quando nel DPEF 2008-2012 proponete per il 2008 una maggiore spesa di 21 miliardi di euro, senza ricorrere ad una manovra correttiva dei conti pubblici, ma soltanto riducendo altre spese di comparto? Anche qui propaganda. Gli italiani, però, vi hanno intercettato e nelle ultime amministrative vi hanno punito severamente sul piano elettorale. Soprattutto al Nord, dove l'economia è più dinamica, hanno capito che questo è il Governo delle tasse, che frena lo sviluppo, rastrella risorse da chi lavora e produce, per distribuirle ai soliti noti: protetti, garantiti, parassiti e clientele elettorali. Avete aperto i mercati dei parrucchieri, dei tassisti, dei farmacisti, per le cooperative della grande distribuzione, ovviamente, ma vi siete ben guardati di aprire i mercati dei pubblici servizi locali, delle tariffe autostradali, dei trasporti pubblici, del mercato dell'elettricità e del gas, delle banche e delle assicurazioni. In questi settori dell'economia italiana, dove non c'è mercato e non c'è concorrenza, perché i servizi siano di qualità e a più basso prezzo, vi guardate bene dal metterci le mani per delle vere liberalizzazioni. Eppure i pensionati, soprattutto quei 10 milioni che vivono con meno di 1.000 euro al mese, quell'11 per cento di famiglie che secondo l'ISTAT vivono in stato di povertà, soffrono la loro condizione di indigenza a causa di affitti alti e tariffe alte per luce, acqua, gas, immondizia e trasporto pubblico. In questo anno di legislatura non avete assunto alcuna misura in questi settori dell'economia italiana, limitandovi a fare elemosine con le tasche di chi paga le tasse. È questa infatti l'opposizione di fondo a questo decreto‑legge n. 81: il modo cioè con cui lo finanziate. Non eccepiamo il merito delle misure, anche se da alcune rimaniamo esterrefatti, come, ad esempio, la norma che sussidia ulteriormente i Comuni confinanti con le Regioni a Statuto speciale per evitare che abbandonino le proprie Regioni di provenienza. Eccepiamo che dette misure si paghino a debito. Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, ha detto con molta chiarezza che il tesoretto non esiste, perché il maggior gettito tributario dev'essere destinato alla riduzione dell'indebitamento. La Commissione europea ha detto, con il commissario Almunia, che le risorse derivanti dal favorevole andamento della finanza pubblica devono essere integralmente destinate al miglioramento dei saldi. Se due autorità indipendenti come Draghi e Almunia, che non sono parte politica, dicono che il bene dell'Italia è la riduzione del debito pubblico, perché il Governo Prodi sceglie di fare la cicala, rinviando il peso dello stesso debito alle future generazioni? Nel DPEF di qualche settimana fa è stato detto che nel 2008 si prevede un rallentamento del commercio mondiale e una riduzione dell'*export* (quest'ultimo straordinariamente favorevole quest'anno). Le misure proposte a favore dei ceti meno abbienti pensioni basse, favoriscono consumi interni che incorporano basso valore aggiunto e perciò favoriscono l'importazione di prodotti elementari, soprattutto afroasiatici. L'aumento dei tassi di interesse della Banca centrale europea indebolisce gli investimenti, rallentando la ripresa. Se questo quadro d'insieme ha una sua validità, irrigidire i conti pubblici con l'aumento della spesa corrente, anche per i prossimi anni, è azione politica grave ed irresponsabile. Questo Governo se ne deve andare prima possibile per il bene dell'Italia! Noi dell'UDC abbiamo proposto un Governo di salute pubblica, ossia un Governo che sostituisca Prodi e si basi su un sostegno parlamentare più ampio, imperniato al centro dello schieramento politico e non più ricattabile da minoranze estreme e radicali. Facciamo appello alle forze più responsabili di questo Parlamento, perché diano vita, prima possibile, a questo Governo di larghe intese, per fare quelle riforme di sistema che servono all'Italia. A Forza Italia e al nascente Partito democratico chiediamo di costruire un altro bipolarismo, dal momento che quello che da quindici anni abbiamo conosciuto non ha consentito di governare, né a Prodi né a Berlusconi. Questa nuova stagione politica che auspichiamo dovrebbe essere sorretta da una riforma elettorale di tipo tedesco, che consenta a ciascuna forza politica di allargare il proprio orizzonte di alleanze in rapporto al tipo di politica che intende sviluppare a favore del Paese e non a favore della coalizione che lo condiziona. Ci si allea non per spartirsi i tesoretti, ma per il bene dell'Italia. Ecco perché siamo contrari a questo decreto‑legge e perché non voteremo mai la fiducia a Prodi, quantunque tra qualche ora essa ci verrà richiesta. Pertanto, l'UDC già in questa fase preannuncia il proprio voto contrario.

assolutamente connotato da falsità sia materiali che ideologiche. Esso è scorretto dal punto di vista politico, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi,

pletora di dispersioni di fondi per venire incontro anche ai movimenti per la lotta all'AIDS, ai Comuni che sono confinanti, come ricordava prima il collega Ciccanti. Si tratta di considerazioni che svolgo non in maniera acrimoniosa, ma fondate su specifiche argomentazioni sia tecniche che politiche. La falsità materiale nel governo della finanza pubblica si è appalesata già con l'insediamento di questo Governo, allorché si decise di affidare alla cosiddetta commissione Faini il compito di certificare i nostri conti pubblici. La scorrettezza di politica economica sta nell'altrettanto evidente circostanza che, in una fase di crescita del Paese, dovuta alle cosiddette esogene internazionali (in altre parole, semplicemente al trascinamento dell'economia internazionale), si preferisce, invece, dilapidare quel tesoretto in mille rivoli di spesa pubblica aggiuntiva, aumentando anche anche le imposte. Tutto ciò avviene, ancora una volta, in dispregio della stessa parola d'ordine - propagandata anche nel DPEF - dello spendere meglio, tanto che in alcune parti il provvedimento provvede a disaccantonare oltre un miliardo di quanto, con baldanza ingiustificata, si era accantonato con la legge finanziaria. Signor Presidente, con noi al Governo le parole d'ordine sarebbero state invece: spendere meno, sprecare meno, soprattutto tassare meno ed investire di più. D'altronde, cosa ci si poteva aspettare da un Governo che ha esordito con il decreto-legge sullo spacchettamento dei Ministeri, un provvedimento ancora oggi non completamente attuato, voluto solamente per regolare i conti della dilaniante lottizzazione, financo dei singoli uffici dei Ministeri? Un Governo che strombazza su presunti interventi sui costi della politica e che, allo stesso tempo, lascia intonse le pletoriche delegazioni all'estero delle Regioni (voglio ricordare quelle della mia Campania, laddove Bassolino ha un ufficio enorme e una serie di consulenti, e ha determinato che la più alta tassa sui rifiuti d'Italia sia pagata da noi campani), gli innumerevoli consigli di amministrazione di enti inutili, le faraoniche spese di enti vari. Ma l'aspetto più grave, secondo noi, è quello della immoralità intrinseca di questo provvedimento. Vedete, nessuno vuole contestare gli aumenti delle pensioni minime, vivaddio, ma è evidente che con pochi euro al mese non si risolverà la situazione di nessun pensionato: al massimo si creeranno aspettative ingiustificate. L'immoralità, ancora, sta nell'aver creato ad arte un tesoretto occultando la maggiori entrate del 2006 e del 2007 2007 dovute sia alla maggiore crescita che al funzionamento dei meccanismi virtuosi dell'ultima nostra finanziaria, quella del centro-destra, del Governo Berlusconi, ed utilizzando poi queste entrate subito per una maggiore spesa. L'immoralità sta in questa ideologia perversa in base alla quale, appena il sistema produttivo crea delle risorse, bisogna subito appropriarsene e dilapidarle in mille rivoli. Questa è l'idea fondante di questo Governo di centro-sinistra, che vede l'imprenditore, colui che produce, come nemico per utilizzare le risorse distribuendole in maniera diversificata. L'immoralità sta nel credere che un Paese che ha il terzo debito pubblico più alto del mondo in valore assoluto possa continuare a scaricare sulle generazioni future l'onere di questo debito, come mettendo la polvere sotto il tappeto e immaginando che le prossime generazioni e i prossimi Governi dovranno L'immoralità sta, ancora, nell'aver adottato questo provvedimento all'inizio di luglio, ad un mese appena dalla pausa estiva, con il preciso calcolo preventivo, quindi, di strozzare e di impedire qualsiasi discussione al Senato, in Assemblea e in Commissione, dato che ci ritroviamo senza relatore e con qualche ora appena di dibattito svolto nella Commissione, nonostante lo sforzo del Presidente e anche probabilmente di qualche collega della maggioranza, con l'intento preciso di vanificare lo sforzo contributivo di miglioramento del provvedimento.

Non poteva esserci una sintesi più efficace per rendere l'idea del momento che stiamo vivendo. Anche sul piano contabile, l'illegittimità giuridica è evidente

1978, non altre; e voi l'avete violata: ecco la vera incostituzionalità

con il ciclo economico. Come più volte raccomandatoci dalle istituzioni europee, il *surplus* di entrate avrebbe dovuto essere utilizzato per ridurre il *deficit*, così da non costringere in un prossimo o immediato futuro, ad effettuare invece una manovra in condizioni di difficoltà. Più rozzamente, ma efficacemente, è stato sostenuto che si stanno avvelenando i pozzi, in danno dei prossimi Governi (del prossimo Governo di centro-destra, come mi

è legata all'attività del Governo precedente: è quindi accaduto esattamente il contrario. Sopravvenienza attiva, cioè, vuol dire che vi è stata una gestione virtuosa della finanza pubblica, che ha creato una crescita dell'avanzo senza aver aumentato le tasse. Ecco

impossibile pagare centinaia, se non migliaia, di euro in più, se è vero quanto avete affermato voi, che avreste ridotto le tasse. Infatti, cos'è accaduto?

velocità nell'andare addirittura contro legge, per tramare l'ennesimo inganno politico, al fine di utilizzare quei soldi che legge italiana non vi consentiva di usare. Ma con questa specie di gioco di *matriosche* state di fatto utilizzando il cosiddetto

prigionieri del partito della spesa. E questo dimostra, come dicevo poc'anzi, che siete assolutamente insicuri: prima dicevate di togliere soldi ai Ministeri e oggi invece date loro 2 miliardi di euro in più, perché è chiaro che sentendo ormai traballare le fondamenta del vostro Governo avete paura di

noi vi poniamo invece dei limiti e soprattutto non vi consentiamo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione. Oggi invece dite: sì, però parte degli avanzi di amministrazione ve li consentiamo e poi vi chiediamo ancora di intervenire nei confronti dell'ICI. Non scendo nei particolari perché credo che qualsiasi comune

le guance rosse, arrossite dal pudore e dall'imbarazzo. In questo decreto c'è una distribuzione a pioggia di soldi per provvedimenti chiaramente clientelari, è stato sottolineato da più parti. Mi colpisce, ad esempio, come ancora una volta si ricorra al meccanismo degli incentivi a pioggia dati alle imprese secondo un vecchio schema, che in realtà nasconde poi logiche di tipo clientelare. Così come mi colpisce una misura anche francamente un po' ridicola, come i sussidi ai Comuni confinanti per evitare che possano passare da una Regione a Statuto ordinario ad una a Statuto speciale. E invece mancano completamente, in questo panorama frammentato e disarticolato, un disegno strategico e interventi strutturali, seri, importanti di cui il Paese ha invece drammaticamente bisogno. In particolare, mancano interventi in due settori veramente importanti, quello dell'università e della ricerca e quello dell'istruzione. Vedete, gli interventi che qui sono previsti in realtà confermano una logica perversa, di tagli e di accantonamenti,

viene mantenuto per gli anni 2008 e 2009, anzi viene definitivamente confermato per tali anni: dunque, per il prossimo anno il mondo della ricerca e dell'università avrà un venti per cento in meno di risorse. Ancora, il discorso degli accantonamenti. Qualcuno ha salutato come una inversione di rotta questo sblocco degli accantonamenti, ma esso interviene soltanto per un terzo. Questo vuol dire che il mondo dell'università non potrà utilizzare centinaia di milioni di euro (risorse significative e importanti) perché accantonate gli altri due terzi che non vengono sbloccati.

Non posso qui non denunciare, per esempio, il fatto che la ricerca italiana è bloccata. Vorrei che in quest'Aula ci fossero in questo momento i senatori Villone e Fisichella, i colleghi universitari che sicuramente hanno a cuore il problema dello sviluppo della ricerca nel nostro Paese. il FIRST, quel grande fondo di investimenti promesso in finanziaria, non è mai stato varato, né è mai stato predisposto un regolamento. Siamo ancora alla logica dei vecchi programmi di che da quando esistono sono sempre stati banditi e pubblicati entro marzo, per consentire ai ricercatori di poter utilizzare questi finanziamenti: ma questi piani di ricerca non sono stati ancora pubblicati e ci avviamo

questo sia un dato drammatico, perché vuol dire che noi, per quest'anno, rischiamo di non poter investire in ricerca. Altro che svolta clamorosa e importante, altro che le promesse fatte nel vostro programma in campagna elettorale con cui avete costruito un consenso politico e che ora, invece, miseramente disperdete! Non posso qui, per esempio, non citare - perché fra l'altro è un illustre personaggio della sinistra italiana - il professor Martinotti, che ha mandato una lettera aperta al ministro Mussi proprio lamentando il fatto che l'università sia ormai alla canna del gas. Ancora, credo che ci siano altri provvedimenti che meriterebbero di essere egualmente considerati nel settore dell'università. Penso, ad esempio, al fatto che avete bloccato l'assunzione dei professori, dei docenti, dei ricercatori

assunzioni. Passando al discorso scuola e istruzione, in realtà, caro ministro Fioroni, come è stato dimostrato da questo provvedimento e da questo dibattito, non vi è alcun buco che il Governo Berlusconi ha lasciato in eredità

quando un professore si ammalava in questo anno scolastico, soprattutto nell'ultima parte, i dirigenti scolastici erano costretti a lasciare i ragazzi a casa o a smistarli nelle altre classi, perché non avevano i soldi, non avevano quei 300 milioni di euro necessari a pagare i supplenti. prevista una piccola reintegrazione, del tutto inadeguata e insufficiente: non lo dico io, l'aveva dichiarato Panini, il segretario generale della CGIL. E, ancora, siete stati costretti, così dire, a ricalcolare, a considerare che avete sbagliato i calcoli della riforma della maturità; avete proposto in quelle norme urgenti (che poi tali evidentemente non avete più considerato, perché sono rimaste alla Commissione bilancio della Camera e chissà quando verranno approvate) di stanziare 51 milioni di euro in più per pagare i commissari di maturità, ma li avete sottratti ai bilanci delle scuole.

ora che continuate a tagliare sui bilanci delle scuole, probabilmente i genitori saranno costretti a portare persino i banchi. Beh, capite, ci troviamo in questa logica di emergenza e per trovare risorse da destinare a spese improrogabili ed inderogabili voi le togliete ai bilanci delle scuole.

disperso a pioggia secondo logiche clientelari e certamente poco produttive, ci saremmo aspettati veramente un cambio di tendenza, come avevate promesso in più occasioni in tutti questi mesi, come in più occasioni l'opposizione e anche la maggioranza avevano in qualche modo invitato il Governo a fare. Nulla di tutto questo è avvenuto: vedo un futuro molto nero per l'istruzione, l'università e la ricerca italiana e quindi un futuro molto nero per il Paese.

onorevoli senatori, con la conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, che da qui a poco vi accingete a votare con l'ennesima fiducia ma col nostro convinto voto contrario, dando ancora una volta un colpo mortale ai conti pubblici e all'economia del Paese. Per esigenze di tempo evito di passare in esame tutte le cifre da voi indicate,

Con un ragionamento a dir poco assurdo e tortuoso del Ministro dell'economia si vorrebbe dimostrare che il grido di allarme del Governo dell'anno scorso era giusto per poter giustificare allora l'aumento indiscriminato e folle dell'imposizione fiscale che ha messo in ginocchio l'Italia e ora invece è altrettanto giusto inneggiare ad un "tesoretto" frutto di un virtuoso programma del Governo per imbrogliare gli italiani illudendoli di un facile aumento di pensioni o di una riduzione del *deficit*, senza però mai parlare di una sostanziale riduzione della pressione fiscale e ridare così slancio all'economia italiana, ormai arretrata in fondo alla classifica dei Paesi europei. dei Paesi europei. Per accontentare solo una certa parte politica estremista della maggioranza è stato imposto ingiustamente agli italiani un fardello pesantissimo di tasse di tutti i tipi, che non solo ha distrutto l'economia, ma ha sfiduciato tutti gli imprenditori, i quali vedono ormai lo Stato soltanto come un padrone schiavista. Con le vostre false manovre finanziarie - più elettorali che finanziarie - e con i vostri falsi in bilancio avete conquistato la disapprovazione di tutte le classi sociali del Paese.

una delle definizioni di predicatori - politici in prima fila - è quella di chi ci rende tristi e ci ridicolizza per il fatto di appartenere al quotidiano di questo mondo, di chi denuncia in modo radicale i comportamenti vigenti e pone risalto alla perfetta fratellanza sociale che perennemente è ostacolata dall'attività dei maligni, sempre pronti a contrastare i buoni propositi di coloro che si sentono di interpretare il mondo in una visione sovrapersonale, ben definita nel termine tedesco "*Weltanschauung*". Il presidente Prodi è una specie di predicatore, che si domanda perché nelle omelie ecclesiali non si parli di tasse e che è costretto a confezionare il suo sermone conformemente ai propositi di un libricino di 281 pagine, di cui conosceva bene i limiti ma che rappresentava lo strumento per contribuire alla vincita delle elezioni, avendovi inserito le condizioni per l'apporto dell'estrema sinistra. Purtroppo, il Presidente del Consiglio, avendo amalgamato una coalizione con all'interno l'utopia dell'estrema radicale, è rimasto prigioniero di una *intellighenzia* che ha elevato quel libricino a vangelo politico e, per la seconda volta in un decennio, ottenuto il Governo della nazione, si comporta in modo ripetitivo. Allora, viene alla memoria un noto epigramma di Marziale, che recita: «Diavolo faceva il dottore, ora si è messo a fare il becchino, quel che fa da becchino faceva già da dottore». In economia è difficile coniugare sviluppo e consumo e quando un Governo è prigioniero del massimalismo unito al pauperismo di una sinistra congelata da esperienze che hanno miseramente fallito laddove applicate, produce un risultato che ha come sostrato il solo elemento persecutorio realizzato con una fiscalità insopportabile, che mal si adatta in un'economia mondiale di mercato. Con il provvedimento al nostro esame si ha la percezione di essere davanti ad una integrazione della pessima legge finanziaria in vigore, con chiari segnali di preannuncio di quella del prossimo anno. L'articolato, gonfiato oltre misura alla Camera recependo anche l'originario Atto Senato n. 1485, appare come una manovra elettorale che distribuisce risorse che non hanno certezza contabile, quindi non esistono, aumentando la spesa pubblica che, considerato i disavanzi delle Regioni in materia sanitaria, porterà nel prossimo anno il rapporto *deficit*-PIL intorno al 3, Eppure nel DPEF l'onorevole Prodi e il Ministro dell'economia hanno dichiarato di voler utilizzare l'extragettito fiscale interamente a riduzione del debito pubblico, così come chiede l'Unione Europea, cui si aggiungono le recenti indicazioni della Banca d'Italia. Ma le opinioni, non sempre rispettabili, cambiano e, ad esempio, dell'extragettito fiscale del 2007, 900 milioni di euro sono spesi per l'incremento dei trattamenti pensionistici di minore importo, con un incremento che in media non supererà i 35 euro lordi e riguarda, quindi, una semplice restituzione del potere di acquisto delle pensioni minime rispetto all'indice inflazionistico dei prezzi al consumo già rilevato nel 2007. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una filosofia di finanza pubblica ispirata alla cura dell'interesse "privato" e non di quello pubblico, come ricorda anche la massima di Platone riportata, forse ironicamente, nella prima pagina del DPEF. Il decreto-legge è un *omnibus* di frettolose e caotiche disposizioni, con misure *una tantum*, senza riforme strutturali e, addirittura, con una delega al Governo per i diritti marittimi, accentua i dubbi di costituzionalità anche in ordine alla recente sentenza della Consulta in materia di decreti-legge e alle considerazioni testé articolate dal senatore Morando, presidente della Commissione bilancio. Un insieme di misure ove spicca l'accordo sulla spartizione del cuneo fiscale a cui parteciperanno banche e assicurazioni con la possibilità di deduzione degli interessi passivi, mettendo sullo stesso piano il sistema industriale con quello finanziario e, con l'allargamento della platea, i benefìci, sebbene minimali, rischiano di essere considerati aiuti di Stato e bocciati a Bruxelles. Per quanto concerne, poi, le *holding* industriali sembra che si stia discutendo del niente a meno che alla norma di legge inesistente non subentrino le ipotesi fatte nei dintorni del Ministero dell'economia. Aggiungiamo, inoltre, che la manovra correttiva della situazione tendenziale per il 2007 è un vero imbroglio se il Governo dovesse convincersi che oggi si siano verificate le condizioni per una manovra espansiva. Sembra che gli andamenti tendenziali della finanza pubblica appaiono appaiono migliori dello scorso anno al punto che il vice Ministro dell'economia è stato in grado di comunicarne non solo la quantità, ma perfino la destinazione. Immediatamente, però, l'annuncio e stato smentito dal ministro Padoa-Schioppa al quale, seppure trasformato in cinico politico da tecnico della finanza prestato alla politica, non sfugge la cristallizzazione del nostro debito pubblico, la cui misura contribuisce a frenare l'economia, creando timori negli investitori esteri sempre più riluttanti a dare fiducia al prodotto di questo Governo. Con tale debito, infatti non esiste "tesoretto" e le maggiori entrate avrebbero dovuto essere destinate al ripianamento del *deficit*; perché se oggi attraversiamo una congiuntura ancora gestibile, è talmente fragile la nostra economia che basta uno scossone, per caso proveniente dai mercati asiatici in sovrasviluppo, per avere un ciclo economico meno favorevole e in grado di metterci in difficoltà rispetto a Paesi più accorti ai loro interessi nazionali. E la Francia ne è un esempio. Infatti chiede all'ECOFIN una dilazione per il ripianamento del PIL nel 2012. Padoa-Schioppa, per l'Italia, si era assunto l'impegno di un aggiustamento strutturale del nostro rapporto *deficit*-PIL di 0.5 punti percentuali per ogni anno dopo il 2007. Con estrema disinvoltura tale impegno, prendendo atto del contenuto del presente decreto, viene smentito con evidente imbarazzo dell'Europa che ha accolto le richieste francesi sulla base di riforme strutturali e abbassamento della pressione fiscale: mentre Padoa-Schioppa ha chiesto la stessa dilazione perché vuole spendere di più, con un piano di risanamento che va a ritroso. Una bella differenza di come vengono valutate le regole dell'economia, quando si deve sottostare all'esigenza di tenere insieme una bislacca alleanza fondata su 281 pagine di promesse elettorali. Gli effetti di quelle promesse sono sotto gli occhi dell'Europa e sulle spalle di noi italiani che abbiamo visto innalzare la pressione fiscale ad indici insopportabili. In tale contesto, la spesa pubblica diventa una variabile indipendente delle sorti del debito pubblico in quanto riferita alle sole entrate. Considerato, poi, che il taglio della spesa previsto dal famoso comma 507 della vigente finanziaria doveva produrre accantonamenti per 5 miliardi di euro nel 2008 e 4,9 miliardi di euro nel 2009 e non essendoci proposta alternativa, non si capisce come si possa affermare che il Governo non adotterà ulteriori manovre correttive con la prossima finanziaria. Sta di fatto che le tasse si impongono per uno scopo ben definito, e a questo serve il riferimento alla disciplina dell'articolo 81 della Costituzione, e se si introita di più rispetto all'obiettivo è ovvio che le somme vadano restituite a chi sono state prelevate, cioè ai contribuenti, o meglio - come chiede Bruxelles - siano utilizzate per ridurre quel Moloch italiano che è il debito pubblico. Anche sull'IRAP si è fatta confusione. Infatti, è stato messo in atto un dispositivo che assomiglia ad una partita di giro, restringendo la percentuale di deducibilità degli interessi passivi ai beneficiari della misura. Non si comprende, inoltre, come funzionano le presunzioni sugli studi di settori e se gli indicatori di normalità economica riguardino una presunzione semplice, grave, precisa e concordante; è inaccettabile in una materia così delicata per le piccole e medie imprese, vessate anche quando, attraverso una sentenza della Corte di giustizia europea, le si vuole favorire restituendo loro l'IVA versata in più per l'acquisto di autovetture ad uso dell'impresa. È prevista una procedura che obbliga professionisti e commercianti a rifare i conteggi più volte, aggravando il peso della pubblica amministrazione sulle aziende che hanno chiuso i conti per il 2006 e sono costrette a ricalcolare nel 2007, in sede di acconto, tutte le auto aziendali per ottenere la riduzione dei costi. Ci aspettavamo di più dall'*intellighenzia* al Governo per la seconda volta e non possiamo fare a meno di prendere atto che l'Italia ha poche possibilità di essere messa in grado di riagganciarsi stabilmente alla ripresa economica soprattutto a causa della pressione fiscale che grava su famiglie ed imprese, prodotta da un Governo che è impotente di fronte alle riforme strutturali, essendo ancora affetto da una persistente sindrome antiberlusconiana che lo rende capace solo di distruggere quello che di buono è stato fatto dal precedente Governo. PRESIDENTE.

Quel "tesoretto" che la maggioranza si appresta a ripartire, in effetti, come ha detto lucidamente Mario Draghi, non esiste. Siamo, infatti, in presenza di un provvedimento che trova la sua copertura sostanziale nell'aumento del *deficit*, in violazione dello spirito, ancor prima che della forma, degli accordi di Maastricht. So bene che il Governo ha presentato una sua ipotesi di copertura, ma lo schema è visibilmente incongruo. L'onere indicato, in termini di saldo netto da finanziare, è pari a 4.131 milioni di euro. una cifra esattamente pari all'extragettito accertato in sede di bilancio di assestamento, ridotto delle maggiori spese, nel frattempo maturate. Sconcerta, innanzi tutto la simmetria delle cifre: 4.131 milioni di miglioramento del saldo, 4.131 milioni di maggiori spese. Si è, quindi, raschiato il fondo del barile, senza alcuna preoccupazione per le eventuali ulteriori spese che, da qui alla fine dell'anno, dovessero maturare. Aggiungo che la spesa effettiva del decreto-legge in termini di indebitamento netto il parametro che vale ai fini di Maastricht - è di gran lunga superiore, pari a 5,6 miliardi di euro. Si dice che la manovra è comunque giusta. Premia istanze sociali che eurocrati, dal cuore di pietra, non riescono nemmeno a concepire. Qui c'è una vistosa contraddizione.

il resto si sparge in una miriade di rivoli. Vogliamo forse discutere, tanto per dire a caso, dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, cui si elargisce un *chip* di 5 milioni di euro? La verità è che le pensioni sono solo una ciliegina sulla torta. La parte più consistente del provvedimento è solo conseguenza del patteggiamento tra le diverse componenti di questa variegata maggioranza. Non ci sarebbe nulla di male, se le risorse fossero sufficienti. Ma la loro inadeguatezza risulta evidente dalla struttura stessa del decreto-legge. La maggior parte delle spese - il 64 per cento del totale - sono coperte solo sul 2007. Tra queste : i contratti di servizio per le imprese pubbliche, gli investimenti per la rete delle Ferrovie dello Stato, dell'ANAS, dell'ENAV e di Poste Italiane. Non ci sembra un criterio razionale. Esso impedisce ogni visione programmatica di medio periodo e costringe ciascuno di questi soggetti a vivere alla giornata. Questo significa che per gli anni successivi si dovrà provvedere con legge finanziaria, dando copertura a quegli 11,3 miliardi di euro previsti dal tendenziale a legislazione vigente, ma non a politiche invariate: terminologia che rischia di occultare una parte della maggiore spesa che non è di carattere discrezionale - per quest'ultima occorreranno altri 10 miliardi - ma è definita e certa ancor prima del varo della prossima legge finanziaria. Tutto ciò dimostra un'indifferenza ai richiami della ragionevolezza e delle compatibilità finanziarie, né si può essere certi che questo sia l'ultimo tributo da pagare. Domani sorgeranno altre necessità e sarà difficile resistere alla tentazione di replicare un pericoloso precedente. Nel DPEF, il Ministro dell'economia aveva enunciato un principio assolutamente condivisibile: «È auspicabile» - è detto nel documento - «che il valore della spesa primaria diventi un punto di riferimento nella discussione parlamentare sul presente Documento di programmazione economico-finanziaria». In sostanza, il Governo chiedeva al Parlamento di rispettare la linea del Piave costituita da un tetto di spesa primaria complessiva di «circa 700 miliardi di euro, pari al 45,3 per All'interno di questo contesto, avrebbero dovuto essere trovate le risorse per finanziare circa 21 miliardi di euro di spesa ulteriore, il che era ed è possibile solo con tagli corrispondenti. L'impostazione, secondo i repubblicani, è corretta. Peccato sia il Governo a disattenderla. Se nel 2007 non si è riusciti a rimodulare la spesa per 5,6 miliardi di euro, come sarà possibile tentare, per il 2008, un'operazione che è quattro volte tanto? Con questo decreto quindi il Governo sta mettendo a dura prova la sua credibilità. Ha dovuto incassare i rimproveri della Commissione europea e francamente inopportuna appare ogni analogia con il caso francese. In quel caso, l'allentamento dei vincoli finanziari è logica conseguenza di una terapia-*shock* volta ad accelerare il ritmo di crescita di quell'economia. Nel caso italiano è solo frutto dell'impotenza decisionale e delle contraddizioni della maggioranza. Ma soprattutto il Governo ha negato le premesse del suo disegno di politica finanziaria per il 2008, ancor prima che la legge finanziaria sia stata presentata in Parlamento. Non riusciamo, pertanto, a comprendere come si potrà far fronte alle nuove esigenze, se non facendo ricorso ad un ulteriore aumento della pressione fiscale: una misura odiosa che ha già suscitato reazioni durissime da parte di tutti i contribuenti onesti che vorrebbero una contropartita adeguata in termini di servizio e prestazioni. Alla fine, il Ministro dell'economia, anche non volendo, come del resto ha fatto finora, sarà costretto a cedere e assecondare questo disegno. È questo il labirinto in cui il Governo si sta cacciando, forse inconsapevolmente, più probabilmente insistendo nel riproporre quella doppiezza culturale, ancor prima che politica, che ne ha finora caratterizzo il respiro. Anche se il fallimento di questa strategia è ormai evidente. La speranza è che le forze ragionevoli della maggioranza facciano al più presto sentire alta e forte la loro voce per arrestare una deriva rovinosa.

svilupperò alcune considerazioni in relazione al disegno di legge che stiamo esaminando e che riguarda l'uso strategico del cosiddetto tesoretto. Nella valutazione del provvedimento all'esame della nostra Assemblea, non possiamo non partire le nostre considerazioni dalle dichiarazioni rese dal governatore della Banca d'Italia Draghi, il quale, nell'audizione di qualche giorno fa, di fronte alle Commissioni congiunte di Camera e Senato, ha testualmente affermato che non esiste un tesoretto da spendere, che la parola tesoretto è fuorviante e che il miglioramento delle entrate (per intenderci: tasse in più che hanno pagato gli italiani) debba essere utilizzato per il risanamento dei conti pubblici. Ricordo altresì che tale impegno era parte integrante della vostra ultima legge finanziaria; vi rammento anche che l'articolo unico, al comma 4, prevedeva che tutti i fondi in più che risultassero da maggiori entrate fiscali dovessero essere utilizzati per il ripianamento del debito. Certo non occorre citare episodi specifici come questo per ricordare la vostra incoerenza, il vostro comportamento ovviamente non costante, tra impegni che prendete e determinazioni che poi assumete. Sempre il Governatore ha ricordato quanto contenuto nel DPEF per il triennio 2008-2011 che, a nostro avviso, avrebbe dovuto essere collegato a questa manovra di spesa pubblica circa la necessità di reperire risorse per interventi correttivi per un ammontare di 11 miliardi di euro, lo 0,7 per cento del PIL, per finanziare impegni già presi da questo Governo e non coperti. Il DPEF prevede altresì che altri 10 miliardi di euro, e sempre nel 2008, debbano servire per alcuni impegni che prevedete di voler assumere e che non avete coperto nello stesso DPEF e, primo caso nell'attività parlamentare, almeno a mia memoria, il DPEF e il Ministro rimandano alla risoluzione parlamentare l'individuazione dei modi per coprire tali maggiori spese che voi prevedete. In altri termini, procediamo alla rovescia: normalmente è il Parlamento che fornisce al Governo indicazioni sulla programmazione, sulla volontà di fornire risposte al Paese, ed il Governo si preoccupa normalmente di reperire le risorse. In questo caso, si agisce al contrario: il Governo fa le promesse ed il Parlamento dovrebbe trovare le risorse per coprire le promesse del Governo. Dal dibattito, signor Presidente, sul provvedimento in esame, è emerso a chiare lettere che con questo decreto-legge siamo tornati indietro di parecchi anni nel modo di legiferare; si tratta proprio dell'esempio classico di come non si dovrebbe legiferare. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una distribuzione di risorse finanziarie aggiuntive di cui non si comprende bene, per la verità, l'effettiva consistenza: si parla di 7,4 miliardi di euro nel 2007 e di circa 100,7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009. Ad una prima analisi, tutto ciò starebbe a dimostrare che la torchiatura fiscale a cui è stato sottoposto il nostro Paese per il combinato disposto di provvedimenti tributari voluti dal vice ministro Visco e dalla legge finanziaria per il 2007 sia stata del tutto eccedente rispetto alle esigenze effettive del risanamento della finanza pubblica, nel senso che siamo andati ben oltre, È evidente che tale eccesso di prelievo fiscale era finalizzato sin dall'inizio a costituire una riserva di risorse da destinare a seconda delle esigenze e delle convenienze politiche nella stessa maggioranza; tale eccesso di prelievo fiscale ha vessato inutilmente i cittadini e le imprese ed ha prodotto l'effetto di rallentare la crescita e lo sviluppo economico. Credo che il Governo, con questa manovra, si stia incamminando su quella che da qualcuno è stata definita (definizione da me condivisa) finanza allegra, quella del cosiddetto *deficit spending*, tentando così di recuperare quel consenso perduto in vista di imminenti scadenze elettorali. In tal modo, però, si pensa solo a danneggiare il Paese e si compie un'opera di miope e piccolo cabotaggio politico, ma la situazione politica della maggioranza attualmente al Governo mi sembra sia proprio questa: da un lato, la volontà di recuperare il consenso, dall'altro, con questo provvedimento, e nel modo in cui questo provvedimento è stato concretizzato, cioè nella distribuzione delle risorse, c'è un richiamo costante di una parte della maggioranza che per rimanere compatta, per consentire e assecondare il volere dell'attuale Governo, chiede delle sicurezze e delle contropartite. Lo stesso dicasi per le organizzazioni sindacali, le quali, nella definizione della distribuzione del cosiddetto tesoretto, hanno, secondo me, avuto un ruolo significativo e importante. L'altro aspetto che mi permetto di sottolineare è relativo ad un tema a me particolarmente caro, quello della spesa sanitaria.

e non sono stati nemmeno coperti tutti. Ma la situazione non è assolutamente cambiata. Il *trend* del *deficit* nel settore sanitario del nostro Paese continua ad essere in crescita. Si parla - così dice la Corte dei conti di circa 6 miliardi di euro per l'anno 2006 e si ipotizza addirittura un disavanzo, sul finanziamento del fondo sanitario del nostro Paese, di circa 9 miliardi di euro

Di fronte a un panorama di questo genere vi siete preoccupati di destinare e di dividere questo cosiddetto tesoretto in modo

che vi apprestiate, non a fare quello che avete annunciato, cioè allentare la pressione fiscale per il prossimo anno, ma, per il panorama che si è creato (e avete perso un'occasione con il tesoretto), ad aumentarla. E questo, per la crescita del nostro Paese, sarebbe veramente un dramma.

è tempo di risarcimento sociale. L'obiettivo del risanamento dei conti pubblici è stato raggiunto, comprimendo però anche i servizi sociali più elementari e i redditi delle fasce più deboli. Oggi parte allora un nuovo cammino. E questo è possibile, non grazie ad artifici contabili, ma a risorse vere, frutto delle scelte e dell'impegno del centro-sinistra. L'extragettito non è eredità del passato Governo, come qualcuno tenta arditamente di sostenere; non è merito di forze che tuttora utilizzano metodi discutibili per mettere in difficoltà e per colpire chi si batte quotidianamente contro l'evasione fiscale; non è merito di coloro che minacciano di rilanciare improbabili disobbedienze in materia di tasse; l'extragettito è il risultato di una equilibrata ed equa politica fiscale, avviata dal Governo dell'Unione. C'è una grande questione culturale, prima ancora che politica nel nostro Paese. Un Governo, moralmente saldo, che non cede alle scorciatoie dei condoni è il più forte argine contro l'evasione e l'elusione fiscale, come dimostra, prima ancora del numero dei controlli promossi dall'Agenzia delle entrate, l'ampliamento della base imponibile. Tra i capisaldi, su cui regge il decreto che stiamo discutendo, ne vorrei evidenziare due: coesione sociale e politiche del sapere, politiche della conoscenza. Queste politiche non rispondono ad una visione di parte, ma all'orientamento che da sette anni innerva l'azione dell'Europa. Questo è il cuore della strategia di Lisbona. Non c'è futuro senza conoscenza; non c'è futuro senza equità. E le due cose devono sempre procedere insieme. L'intervento a favore dei pensionati più deboli, che vengono con il provvedimento in esame parzialmente risarciti era atteso ed auspicato. La misura è parziale, ma non lo è il principio politico che lo ispira, quello di operare sempre ogni sforzo possibile per garantire dignità a chi ha lavorato una vita. Non deve passare poi sotto silenzio lo sblocco di più di 600 milioni di euro a favore dei comparti del sapere. Queste risorse saranno restituite alla scuola, all'università, alla ricerca ed alla cultura. Dagli stanziamenti per gli enti di ricerca all'edilizia universitaria, dallo sblocco del fondo per l'innovazione fino alle borse di studio per i dottorandi, dall'aumento del FUS al giusto reddito per i precari della scuola, sono diversi gli investimenti previsti in uno dei campi che più erano stati sacrificati dall'intervento di risanamento. A questi settori strategici per la crescita del Paese e per la coesione sociale la finanziaria 2008 dovrà continuare a prestare attenzione. Rivendica tale impegno il fatto che abbiamo i tassi di laureati tra i più bassi d'Europa, soprattutto nelle materie scientifiche e tecnologiche, che il nostro sistema produttivo investe poco e male nella ricerca, che i nostri ricercatori e dottorandi sono pagati la metà dei colleghi europei, che ancora scontiamo, anche nella scuola, il profondo divario tra Nord e Sud. Affrontare questi ritardi è una indicazione netta e precisa del DPEF appena approvato. Esso ha segnato il cammino di cui questo decreto - che stiamo esaminando - è il primo passo.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, siamo chiamati oggi a discutere un provvedimento complesso, che contiene una lunga serie di interventi di spesa, senza alcun criterio organico e senza alcuna logica che guidi la necessità di effettuare queste spese. Il decreto-legge, infatti, mette insieme misure attinenti alle materie più disparate, dai fondi per le pensioni minime a quelli per le missioni di pace, a quelli per i giovani, alla correzione per le rendite dei terreni agricoli alla proroga di smaltimento dei rifiuti elettronici ed ad una delega al Governo per i diritti marittimi. Si tratta per lo più di misure di breve respiro, slegate l'una dall'altra, senza alcuna traccia di riforme strutturali, che sarebbero invece necessarie sopratutto per rimodulare il sistema degli ammortizzatori sociali. Vi sono, invece, solo misure *una tantum*, come quelle finalizzate ad innalzare le pensioni minime ed una miriade di nuove spese: dalla politica di rigore estremo tesa a destinare tutto l'extragettito al ripianamento dei *deficit* di bilancio, si è passati alla politica della spesa allegra, cedendo alle pretese della sinistra estrema. La valutazione del provvedimento in esame deve, infatti, essere inserita nel contesto generale dell'andamento dei conti pubblici ed in tale contesto si pongono diversi interrogativi, primo fra tutti se effettivamente siamo in condizione di spendere risorse aggiuntive derivante dall'extragettito fiscale piuttosto che utilizzarle per diminuire il debito, obiettivo primario imposto dagli impegni assunti con l'Unione Europea. La risposta è decisamente "no". L'Italia non può permettersi un'ulteriore espansione della spesa e questo perché non ci sono dati certi e verificabili sulla strutturalità dell'andamento positivo delle entrate e quindi non sappiamo quanto derivi dalla crescita e dallo sviluppo e quanto sia dovuto alla lotta all'evasione fiscale. Non possiamo quindi prevedere se tali effetti saranno duraturi nel tempo e non siano invece di natura congiunturale. Ma il quesito che ci poniamo è: se se l'andamento delle entrate è così tranquillizzante, perché rimandare l'attuazione del piano di rientro del debito e il conseguimento del pareggio di bilancio, obiettivo così importante per i Paesi della zona dell'euro? Il secondo interrogativo che l'UDC pone è se sia giusto spendere in questo momento. Anche in questo caso, la risposta è che adottare provvedimenti di spesa al di fuori del quadro complessivo delle entrate e delle uscite fornito dalla legge finanziaria è poco responsabile, perché rischia di alterare tale quadro e di rendere necessari degli interventi correttivi. Infine, sorge l'interrogativo se sia giusto spendere così e anche qui noi dell'UDC contestiamo questo metodo, figlio della logica della spesa pubblica spinta dalle entrate fiscali. In questo modo si innesca un meccanismo perverso per cui tutte le entrate derivanti dalle tasse provocano l'espansione della spesa, e più si spende più si è costretti ad alzare la pressione fiscale. In tale contesto, la spesa pubblica diventa una variabile indipendente dal livello del debito pubblico, essendo legata appunto solo alle entrate. Non riteniamo giusto spendere in questo modo, anche in considerazione di una legge finanziaria come quella dello scorso anno incentrata su un aumento delle spese finanziato con l'aumento delle entrate. Questo provvedimento, in ultima analisi, rappresenta il fallimento della parte della legge finanziaria per il 2007 che prevedeva tagli di spesa: tutte le misure relative ai tagli di spesa e alla riorganizzazione della pubblica amministrazione sono risultate inattuate. In particolare, l'articolo 7 di questo decreto è la certificazione del fallimento del taglio lineare previsto dal comma 507 della finanziaria, ciò a testimonianza del fatto che tale tipo di tagli indiscriminati sono il metodo sbagliato per contenere la spesa pubblica, perché vanno nella direzione opposta rispetto alla necessità di razionalizzare e rendere efficiente la spesa, ovvero di tagliare laddove necessario, convogliando invece le risorse dove effettivamente servono. Ricordo che l'UDC, in occasione della discussione della scorsa legge finanziaria, sia in Commissione che in Aula, ha insistito a lungo sulla necessità di modificare il criterio di taglio delle spese così come stabilito dal comma 507; oggi il Governo è costretto a riconoscere che quella critica era ampiamente fondata. L'unico intervento che giudichiamo opportuno è quello relativo all'aumento delle pensioni minime, previsto dall'articolo 5, sul quale però il Governo dovrebbe intervenire al fine di evitare che gli aumenti riguardino anche quelle pensioni minime che però sono inserite in un contesto di redditi familiari ricchi. Ad esclusione di questa misura, doverosa nei confronti delle tante persone anziane, cui è necessario assicurare una pensione che permetta loro un'esistenza dignitosa, tutte le altre non corrispondono a un disegno organico di riorganizzazione della spesa e contraddicono al criterio di responsabilità, di efficienza e di efficacia, continuando a seguire l'impostazione di una pubblica amministrazione vista più come ammortizzatore sociale che come fattore di sviluppo economico. Giudichiamo poi del tutto insufficiente l'impegno del Governo diretto ad attenuare l'impatto degli studi di settore sul lavoro autonomo e sulle piccole e medie imprese, sollecitato non solo dalla giusta protesta delle categorie interessate,

In ragione di tutte queste considerazioni, l'UDC ha adottato la scelta di presentare quasi tutti emendamenti soppressivi delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, di cui si contesta sia il metodo, che il contenuto. Purtroppo, la fase emendativa sarà inutile perché, se il Governo porrà la questione di fiducia, gli emendamenti non avranno accoglimento e attenzione. Purtroppo, dobbiamo constatare che anche il DPEF è figlio di quella politica economica irresponsabile rispetto alla spesa e poco lungimirante rispetto agli obiettivi, poiché elenca una serie di interventi, anche molto ambiziosi, senza però prestare la dovuta attenzione alle risorse necessarie per attuarli. Temiamo che, proprio a seguito dell'espansione della spesa e del cattivo utilizzo delle risorse disponibili, saranno necessarie manovre correttive, nonostante le previsioni ottimistiche del Governo. In conclusione, vorrei ribadire la posizione fortemente critica dell'UDC su questo provvedimento, espressione di una politica economica adottata da questo Governo, che non sostiene la crescita, non incentiva lo sviluppo e non soddisfa le reali esigenze del Paese.